signori Ministri, senatrici e senatori, la Nota di aggiornamento del DEF rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del Paese: alla Nota di aggiornamento risultano allegate le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. È altresì annessa la Relazione al Parlamento (di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale. Lo scenario macroeconomico internazionale illustrato nella Nota evidenzia una crescita dell'economia nel 2018 meno diffusa e solida di quanto ipotizzato nel DEF dello scorso aprile: nella prima metà del 2018, infatti, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno, con rallentamenti in alcune economie avanzate e prospettive di crescita disomogenee tra le economie

soprattutto in relazione alle crescenti tendenze protezionistiche derivanti principalmente dalle politiche dell'amministrazione statunitense. Elevati restano anche altri fattori di rischio globale, come la volatilità delle quotazioni del petrolio e l'incertezza relativa alla Brexit. Per quanto attiene specificamente all'Italia, nella prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3 per cento nel primo trimestre e in decelerazione allo 0,2 per cento nel secondo trimestre. Il rallentamento della crescita è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017. Di conseguenza, il prodotto interno lordo in termini reali non ha ancora recuperato il livello pre-crisi. La Nota di aggiornamento presenta quindi le previsioni aggiornate della finanza pubblica a legislazione vigente per il periodo 2018-2021, che indicano un rialzo della stima annua di indebitamento netto rispetto al DEF dello scorso aprile per tutti gli esercizi considerati. Lo scenario tendenziale prefigura una crescita del PIL pari allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 per cento sia nel 2020 che nel 2021. In particolare, per l'esercizio in corso, la previsione di indebitamento netto in rapporto al PIL, sia pure in calo sul precedente anno, registra un peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, attestandosi all'1,8 La revisione delle stime comporta un peggioramento dei valori attesi del saldo anche per gli esercizi 2019-2021: dallo 0,8 per cento all' 1,2 per cento per il 2019, da una previsione di pareggio a un disavanzo dello 0,7 per cento per il 2020, da un avanzo dello 0,2 per cento a un disavanzo dello 0,5 per cento Alla revisione del saldo di indebitamento netto, rispetto al precedente quadro tendenziale, contribuiscono sia l'andamento dell'avanzo primario sia la spesa per interessi. Complessivamente, nelle nuove previsioni, l'avanzo primario in rapporto al PIL conserva un profilo di crescita, ma meno accentuato rispetto al DEF di aprile, attestandosi al 2,4 per cento nel 2019, al 3 per cento nel 2020 e al 3,3 per cento nel 2021. La Nota di aggiornamento 2018 aggiorna quindi il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-2021. Gli obiettivi di saldo netto da finanziare (SNF) programmatico del bilancio dello Stato in termini di competenza sono stabiliti nel limite massimo di 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020, e 45,5 miliardi nel 2021. Nella relazione al Parlamento, il Governo illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, che per l'Italia coincide con il pareggio di bilancio strutturale. Nello specifico, annuncia che il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine riprenderà solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare, quando il tasso di disoccupazione e il PIL *pro capite* in termini reali saranno tornati ai livelli pre-crisi. L'obiettivo programmatico di indebitamento netto è fissato quindi al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante a meno 1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Tale percorso viene giustificato da un incompleto recupero dei livelli di reddito procapite rispetto ai valori pre-crisi, da persistenti squilibri territoriali, dalla revisione al ribasso della crescita effettiva nel primo semestre del 2018, dal deterioramento delle prospettive macroeconomiche internazionali, dal deprezzamento del tasso di cambio dei concorrenti internazionali, da previsioni al rialzo del prezzo dell'energia e del petrolio in particolare. I tassi di crescita delineati nel quadro tendenziale a legislazione vigente sono ritenuti dal Governo inaccettabilmente bassi, così come quelli che deriverebbero dal perseguimento alla lettera degli obiettivi di indebitamento previsti dalle regole europee. Il Governo ritiene, infatti, che una politica di bilancio restrittiva priverebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo, nonché la sostenibilità sociale. Quest'orientamento è supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale e dell'*output gap*. La Nota chiarisce inoltre che le maggiori risorse finanziarie rese disponibili dalla revisione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine verranno destinate, in primo luogo, a sostenere la crescita attraverso il rilancio e il potenziamento degli investimenti pubblici e privati, allo scopo anche di ridurre i divari territoriali. Verranno effettuati maggiori investimenti pubblici, consistenti in particolare in un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana: inoltre il Governo intende favorire la ripresa di tali investimenti tramite la messa a punto di una *task force* per migliorare la capacità delle amministrazioni pubbliche di preparare, valutare e gestire piani e progetti. Altro strumento per la ripresa degli investimenti sarà il coinvolgimento delle società partecipate o titolari di concessioni pubbliche. Per quel che riguarda, invece, gli investimenti privati, solo un credibile e prolungato sostegno ai redditi, secondo il Governo, può migliorare le aspettative delle imprese e portare a una più decisa ripresa dell'accumulazione. Con lo scopo, quindi, di migliorare tali aspettative, oltre che con quello di migliorare l'inclusione sociale e incentivare il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro (anche allo scopo di potenziare le competenze necessarie all'innovazione), il Governo intende adottare due ambiziosi provvedimenti. Il primo è il reddito di cittadinanza, che ha in primo luogo lo scopo di aumentare la mobilità del lavoro, incentivando l'accumulazione di capitale umano attraverso la formazione della forza lavoro e l'adattamento delle capacità dei lavoratori a quelle richieste dai rapidi cambiamenti tecnologici, che cambiano le esigenze del mercato del lavoro. Ciò avverrà attraverso la ristrutturazione e il potenziamento dei Centri per l'impiego. In secondo luogo, il reddito di cittadinanza andrà a contribuire al miglioramento della qualità della vita delle tante persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e relativa. Il secondo provvedimento consiste nel superamento della cosiddetta legge Fornero e nell'introduzione di forme di pensionamento anticipato. Ciò permetterebbe ai lavoratori anziani di andare prima in pensione e, contemporaneamente, favorirebbe il ricambio generazionale e l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Tale ricambio è fondamentale nell'ambito della transizione verso la cosiddetta Impresa 4.0, ovverosia il processo che porterà ad una produzione industriale sempre più automatizzata e interconnessa. Affinché il nostro Paese sia preparato a questo passaggio, è vitale che i giovani possano portare nel mondo del lavoro le conoscenze acquisite durante gli anni della loro formazione. La Nota riferisce inoltre che gli aumenti di IVA e accise previste per il 2020 e 2021 verranno «parzialmente» neutralizzati, rinviandone ai prossimi esercizi finanziari la cancellazione completa. Quanto infine al debito pubblico, nella Nota il Governo dichiara di condividere l'obiettivo di riduzione del rapporto debito-PIL, pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia rappresentato dall'aumento del denominatore risultante da un'accelerazione della crescita economica favorita dalla manutenzione del territorio e delle infrastrutture e dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche in capitale umano e innovazione. Un'azione sul numeratore del rapporto attraverso una restrizione di bilancio, invece, potrebbe mettere a rischio, nella visione del Governo, la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commercio internazionale, di elevato tasso di disoccupazione - soprattutto giovanile - e di ridotti investimenti. Nello scenario programmatico, quindi, come conseguenza dei provvedimenti che il Governo intende adottare, la Nota profila un tasso di crescita del PIL dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021. Tale maggior crescita contribuirà al miglioramento degli indicatori relativi al rapporto debito-PIL. Nella Nota, infatti, si prevede per l'anno in corso una riduzione del rapporto debito-PIL al 130,9 per cento, determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5 per cento) superiore alla crescita dello *stock* di debito (2,3 La riduzione del rapporto debito-PIL appare ancora più marcata nel percorso programmatico fissato dal Governo per il triennio 2019-2021, nonostante il livello dello *stock* di debito presenti un andamento crescente di anno in anno.

Per quanto riguarda la regola del debito prevista dalla *governance* economica europea e recepita nell'ordinamento nazionale con la legge n. 243 del 2012, la Nota indica che il valore di riferimento non verrebbe conseguito nella versione prospettica sia nel 2018, sia nel 2019, con un divario compreso tra il 3,1 e il 4,2 per cento del PIL per il 2018 tra il 2,4 e il 3,9 per cento per il 2019, a seconda che si consideri lo scenario tendenziale o quello programmatico. Il Governo pone tuttavia in evidenza come i fattori rilevanti che caratterizzano l'attuale congiuntura economica verranno necessariamente presi nella dovuta considerazione dalla Commissione europea nel valutare il rispetto della regola.

da solidi fondamentali dell'economia e della finanza pubblica italiana. La proposta di politica di bilancio del Governo appare equilibrata e caratterizzata da caute ipotesi sugli effetti che le misure potranno produrre sulla crescita. Il Ministro ha rilevato inoltre che, a differenza di quanto ipotizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), il moltiplicatore delle misure diverse dalla disattivazione della clausola di salvaguardia risulta ben inferiore all'unità, e quindi compatibile con le principali risultanze scientifiche in materia e del tutto in linea con quello ottenuto dai principali modelli in uso nelle istituzioni internazionali. Quanto alla tempistica delle misure, nella consapevolezza della necessità di attivare quanto prima gli investimenti e le misure di inclusione sociale previste per la tenuta del tessuto economico-sociale, il Governo ha interpretato le obiezioni dell'UPB come uno stimolo all'azione anziché un motivo per rivedere verso il basso le proprie previsioni e le proprie ambizioni. Il Ministro ha quindi concluso con un richiamo alla necessità di un quadro di pieno coordinamento istituzionale, evidenziando che gli interventi proposti si muovono nell'ambito degli strumenti messi a disposizione dalla *governance* economica europea per permettere ai Paesi membri di meglio adattare le proprie politiche ai mutati contesti macroeconomici. intendo sottolineare che la Nota di aggiornamento si pone come obiettivi principali la crescita, la buona occupazione, la ripresa degli investimenti pubblici e privati, il rilancio della ricerca, la promozione dei settori chiave dell'economia (*in primis* il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni) e, soprattutto, la lotta a tutte le forme di povertà che colpiscono in misura sempre maggiore non solo i disoccupati, ma anche i lavoratori e i pensionati. Tutto ciò, naturalmente, deve avvenire senza trascurare la tenuta dei conti pubblici. Riteniamo che la crescita e la disciplina di bilancio possano coesistere e la Nota di aggiornamento presenta un percorso di riduzione del *deficit* che non sacrifica la crescita ma che, anzi, trae giovamento da questa. Quella che si svilupperà nei prossimi mesi sarà la prima manovra di bilancio di questo Governo. I miglioramenti che ne deriveranno per la qualità della vita, per gli indicatori di *performance* e per quelli di sostenibilità del debito pubblico metteranno in evidenza la bontà delle nostre scelte e ci spingeranno, nei prossimi anni, a fare ancora di più per le fasce più deboli della popolazione, per i giovani e per l'impresa. I nostri pareri potranno divergere sulle scelte che il Governo compie e sulla bontà delle linee di intervento, ma io credo che il dibattito si debba concentrare sull'opportunità di compiere una scelta di politica economica di carattere espansivo, sicuramente ambiziosa, ma che non fa venir meno l'obiettivo di medio termine, lo rimodula e cerca di aumentare - riuscendoci, nel quadro programmatico

del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo. Ai sensi del richiamato articolo 6, commi 3 e 5, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta; il secondo, relativo alla Nota di aggiornamento, da votare a maggioranza semplice. Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la fine della discussione. Dichiaro aperta la discussione.

ho ascoltato con attenzione la relazione; speravo potessero emergere nuovi elementi, vista la serie di giudizi serie di giudizi negativi che sono stati espressi in questi giorni, ma anche i suggerimenti che provenivano da altre forze politiche. Purtroppo così non è stato:

ritrovarci insieme per sostenere i princìpi che fino ad ora ci hanno contraddistinto. Ero già intervenuto in occasione sul DEF per parlare di un settore che, anche dalla relazione, mi sembra trascurato: mi riferisco all'agricoltura, che tra l'altro investe gran parte dei nostri lavoratori sui territori.

leggo testualmente - di semplificazione delle procedure da estendersi a tutti i settori produttivi; riduzione degli oneri burocratici; istituzione di un patto per la semplificazione in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'indicazione dei risultati attesi e dei tempi; riorganizzazione del Ministero; tutela del *made in Italy* agroalimentare per contrastare la contraffazione e rendere la produzione più sostenibile. Ho citato testualmente, perché sembrano veramente frasi uscite fuori dal tubolario di vecchia memoria, vista l'inconsistenza. E così si può andare avanti: protezione delle indicazioni geografiche nel mondo e sul *web* e contrasto all'*italian sounding*; azioni di *marketing* territoriali e resa operativa dei distretti del cibo, con la creazione di un apposito registro nazionale. Potrei continuare ancora per molto, però, colleghi, quello che mi preoccupa è che non si parla né di modi né di tempi. Abbiamo provato anche in Commissione a dare non solo come minoranza, ma anche dalla maggioranza sono venute indicazioni in merito a tematiche quali l'introduzione di sgravi fiscali, la riduzione - a partire da subito - dei costi energetici per la produzione agricola. tutti i nostri appelli sono caduti nel vuoto. Questa situazione ci preoccupa molto e non ci fa ben sperare. di aggiornamento ci sono molti proclami e buone intenzioni. Come recita un famoso detto, di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno. Mi auguro che non sia questo il caso, né per gli italiani né per l'Italia, perché si meritano molto altro e molto di più di quanto che c'è scritto in questa Nota.

Signor Presidente, componenti del Governo, pregiatissimi onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che ci accingiamo a discutere e approvare rispecchia gli orientamenti e le strategie di quel Governo, definito «del cambiamento», che legittimamente è stato eletto e voluto dai cittadini italiani, dopo tanti anni di Governi tecnici o nominati *ad personam*. In questo momento di democratico e proficuo confronto in Assemblea, ritengo però utile e opportuno approfondire uno dei temi fondamentali dai quali il Governo del cambiamento non potrà prescindere, ovvero la ricerca e le professionalità coinvolte. Le politiche adottate negli ultimi vent'anni in tema di formazione *post*-scolastica ci hanno restituito un Paese inospitale nei confronti della ricerca e delle sue professionalità. un sistema universitario che, a confronto con quello degli altri Paesi europei, appare agonizzante, profondamente iniquo e per nulla attrattivo. È agonizzante perché costantemente definanziato, sottodimensionato e sempre più vecchio. Nel confronto internazionale, invero, l'Italia si colloca al quindicesimo posto rispetto ai venti Paesi OCSE, con una spesa per ricerca e sviluppo ferma

Nel 2017, le risorse destinate a tale fondo sono rimaste sostanzialmente costanti. Stessa situazione si ha con riferimento al personale impiegato in ricerca e sviluppo, che si attesta al 10 per cento dell'intera forza lavoro, contro un valore medio europeo pari al 13 per cento. Notevolmente inferiore è anche la quota di ricercatori rispetto al totale del personale impiegato in ricerca e sviluppo, pari al 48,3 per cento, contro una media europea del 63,4

Francia, il 43 della Germania e il 34 dell'Olanda. Nel nostro Paese si accede al ruolo di ricercatori alla soglia dei quarant'anni e l'età media dei ricercatori supera i In aggiunta, l'attuale sistema pubblico della ricerca genera diseguaglianze, poiché non favorisce pari opportunità, tanto a livello territoriale, quanto sul piano della dignità professionale di quanti vi operano. Sul piano territoriale, i dati Istat sulla spesa e sul personale impiegato in ricerca e sviluppo restituiscono un ampio e allarmante divario tra le Regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. Mentre le prime presentano valori di spesa e di personale pressoché allineati a quelli europei, le Regioni meridionali si posizionano Il sistema che ereditiamo, dunque, salva pochi poli di eccellenza al Centro-Nord, mettendo in crisi la gran parte delle università e degli enti di ricerca al Sud, con il rischio di privare tali territori ed i collegati ecosistemi economici di importanti opportunità in termini di qualificazione del capitale umano, innovazione e, più in generale, di sviluppo socio-economico. A ciò si aggiungono gli effetti perversi che l'attuale sistema di reclutamento del personale docente e ricercatore ha generato negli ultimi dieci anni in termini di precariato, privilegi, blocco delle progressioni di carriera e del *turnover*. avvenuto in un clima di profonda conflittualità tra le diverse figure universitarie, ormai di dominio pubblico e oggetto di contenziosi e azioni collettive di tutela dei diritti costituzionalmente negati. Emblematica è, in tal senso, la posizione dei ricercatori universitari: al 1° gennaio 2018 i ricercatori in organico alle università italiane sono 19.277; di questi 13.900 sono ricercatori a tempo indeterminato 2.322 sono ricercatori precari privilegiati. Il quadro delineato evidenzia un Paese per nulla attrattivo non solo per i ricercatori italiani, ma anche per quelli stranieri, che reputano evidentemente più vantaggiosi e stimolanti altri contesti europei. Il sistema della ricerca quindi, data la situazione in cui versa e considerata l'importanza strategica che riveste per la crescita e la competitività del Paese, necessita di un piano strategico di rilancio che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che attualmente lo caratterizzano e ne frenano le sue prospettive di sviluppo. Sono queste le condizioni necessarie per non perdere e attrarre quel capitale umano necessario per sostenere e valorizzare l'innovazione tecnologica indispensabile per il raggiungimento degli auspicati obiettivi di crescita economica. Non ci può essere vero cambiamento economico, sociale e culturale senza un adeguato sistema di ricerca.

Signor Presidente, ho letto molto attentamente e con molto interesse la Nota di aggiornamento al DEF e ho visto anche oggi tanti iscritti a parlare che analizzeranno in modo dettagliato

quindi, non è decisivo in tal senso, ma non è accettabile per noi che le autonomie speciali non vengano trattate e vengano lasciate da parte. Come rappresentante delle autonomie speciali delle minoranze linguistiche, spero che nei provvedimenti che seguiranno a questa Nota di aggiornamento venga data la giusta attenzione alla nostra specificità. Nella Nota di aggiornamento si parla di riforma costituzionale, ma non vi è un solo cenno alla tutela e valorizzazione delle autonomie. Lo stesso è accaduto anche con il contratto di Governo e nel primo discorso che il Presidente Conte ha svolto in questa Aula.

Signor Presidente, componenti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la Nota di aggiornamento al DEF è il primo vero atto di programmazione economica e di indirizzo politico di questo Governo. ultimi giorni, nella Commissione bilancio di cui faccio parte si sono susseguiti in audizione organismi indipendenti che hanno il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. La partita si è giocata su complessi calcoli statistici e modelli econometrici che, nella maggior parte dei casi, hanno invitato alla prudenza o espresso preoccupazioni. In realtà, veniamo da anni difficili, da manovre repressive, da quella austerità in cui siamo precipitati nel 2011 e dalla quale non siamo riusciti a rialzarci nonostante il *trend* positivo internazionale

compaesana, che hanno mandato nello sconforto tanti concittadini che avevano l'aspettativa di godersi finalmente il meritato riposo dopo anni di lavoro, e cito l'esempio più eclatante. Quelle manovre restrittive non hanno fatto altro, però, che provocare una contrazione dell'economia italiana: le aziende più importanti sono fuggite dall'Italia e chi è rimasto ha incontrato tempi duri. Il risultato di tutto questo sacrificio qual è stato? un PIL reale che, dopo anni di segno negativo, ha cominciato timidamente a crescere trainato esclusivamente dalla congiuntura positiva internazionale. Il debito pubblico è aumentato fino a toccare il 132 per È allora evidente che, seppur i calcoli siano complessi, qualcosa non è andato per il verso giusto, perché qui si parla di previsioni, di scenari possibili. I conti sul futuro non si fanno con numeri certi, ma con numeri che hanno un certo livello di confidenza dietro i numeri ci sono delle ipotesi. È quindi evidente che la rigidità dei modelli econometrici ha portato a previsioni sbagliate, ma

Le indicazioni contenute nel DEF rispecchiano ciò che gli italiani si aspettano da questo Governo e da questa maggioranza parlamentare. La manovra annunciata dal DEF sarà finalmente espansiva e andrà finalmente ad agire sul denominatore di quel rapporto fatidico debito/PIL debito/PIL per cui tanto ci giudica l'Europa. È ovvio: bisogna essere realisti che questo è un inizio. Centinaia di migliaia di lavoratori bloccati dalla Fornero potranno finalmente scegliere di andare in pensione; la *flat tax* interesserà inizialmente le partite IVA e le piccole attività; l'incentivo sarà riconosciuto anche alle aziende soggette all'IRES che investono nel futuro. Ci sono poi lo sblocco degli investimenti pubblici, la semplificazione delle procedure, tutte misure espansive. Non sto comunque a dilungarmi dopo l'esaustiva relazione del collega Dell'Olio. Ieri nella discussione generale in Commissione - peraltro da me molto apprezzata l'ammissione è stata generalizzata, se non ho capito male anche da parte delle opposizioni: la strategia è certamente da cambiare e, quindi, occorre agire sul denominatore del rapporto debito/PIL. Ebbene, sappiamo tutti che questo nostro cambio di rotta sarà sotto la lente di ingrandimento dell'Europa; i Governi europei ci osservano, così come i popoli europei. Il rischio di turbolenze dei mercati non ci spaventa. Sono dell'idea che non si comanda un popolo a botte di *spread*.

la Nota di aggiornamento al DEF 2018 conferma tutti gli impegni più popolari presi in campagna elettorale da Movimento 5 Stelle e Lega, ma è evidente che per la sanità nella prima legge di bilancio giallo-verde il triennio 2019-2021 segna il buio pesto. Unica ragionevole certezza è che il miliardo aggiuntivo stanziato dal precedente Esecutivo rimarrà indenne, con un finanziamento pubblico per il 2019 di 114,396 miliardi.

Invece, nonostante l'aumento del debito pubblico, tutela della salute, ricerca, sviluppo e innovazione non hanno diritto di cittadinanza nella manovra di fine anno. Questo Documento azzarda una crescita del PIL del 3,1 per cento nel 2019, del 3,5 nel 2020 - e tutti ce lo auguriamo - ma prevede il rapporto PIL/spesa sanitaria al 6,4. Vorrei ricordare che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, quando questo rapporto scende sotto il 6,5 per cento, si mette gravemente a rischio l'erogazione dei servizi. tutto questo è nettamente in contrasto con le parole pronunciate dal *premier* Conte quando si è presentato a chiedere la fiducia alle Camere, dicendo che la sanità era la priorità in cima al programma di Governo: non mi sembra. Il ministro Grillo il 2 agosto in audizione ha detto che avrebbero aperto i rubinetti: mi sembra che i rubinetti siano stati aperti per altro

ma il Governo ha già confermato il via libera al regionalismo differenziato, che - come sappiamo tutti - aumenterà le disuguaglianze. Si propone di aumentare l'attenzione per la promozione e la prevenzione della salute senza prevedere azioni correlate, né tantomeno risorse; non si considera il rinnovo delle tecnologie e la formazione del personale. A proposito di rinnovo dei contratti del personale, è stato calcolato che solo quello del personale medico e paramedico costerà circa un miliardo,

Non parliamo del *payback*: non c'è un conteggio e le aziende devono sapere cosa accantonare ma non se ne parla. Riguardo a promozione, innovazione e ricerca vedremo come riusciremo a implementare il fascicolo sanitario elettronico.

Per l'investimento nel patrimonio edilizio sanitario servirebbero, secondo la Corte dei conti, 32 miliardi. Pertanto, ci sono poca chiarezza e scarsi numeri; nessun riferimento alle politiche su famiglia, natalità, disabilità; nessuna parola sul *caregiver;* non si fa riferimento al fondo per i farmaci innovativi, innovativi, né alle coperture. Sul numero chiuso il Ministro ha di nuovo cambiato idea: certo che lo si può togliere, ma deve essere concretizzato un investimento, perché gli studenti devono poter avere aule che non ci sono. Quindi, prima di parlare è meglio fare i conti, e anche prima di presentare conti fasulli. fasulli. Manca totalmente un approccio per salvare il Sistema sanitario nazionale; le azioni innovative sono poche; non c'è un programma; non c'è una programmazione reale per i prossimi cinque anni e non ci sono investimenti. Io sono molto preoccupata, ma sembra essere chiaro che la sanità al momento non rappresenta una priorità né per Di Maio né per Salvini. *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, signori rappresentanti del Governo, finalmente in Aula, dopo la fase degli annunci, dopo le audizioni e gli scontri su scenari macroeconomici ipotetici, dopo la Commissione, dove ho cercato di spiegare, con dovizia di particolari, quello che adesso dirò in qualche minuto. Finalmente l'Aula, per ragionare di fatti. i fatti sono che l'Italia in questo momento perde peso, credibilità, ricchezza. I fatti, che non sono belli, ma sono oggettivi, ci parlano di uno *spread* che cresce e di vendite a pioggia in Borsa, che si stanno mangiando, già prima, la cosiddetta manovra del popolo. Dal 26 settembre, quando è stato annunciato il *deficit* al 2,4 per cento - quando invece il 17 settembre 17 settembre proprio il ministro Tria aveva garantito sull'1,6 per cento - la curva dei rendimenti dei BTP è tornata ai livelli del 2013; il costo delle polizze contro il rischio *default* dell'Italia è tornato ai tempi di maggio, al momento della crisi (quando non si capiva quale sarebbe stato il futuro del Paese); il costo delle parole - il *copyright* non è mio, ma è del presidente della BCE Draghi - è stato pari all'aumento di 2 miliardi di euro della spesa per interessi, come viene riconosciuto nella stessa NADEF. Potrei parlare di molte cose. Non voglio parlare del reddito di cittadinanza; dico soltanto che non tornano i conti, perché 780 euro per 6,5 milioni di persone fa 50,7 miliardi e non 10 miliardi. Naturalmente questo ci fa pensare che verrà inserita una serie di limiti che farà sì che venga annullata la questione in sé. contro le spese immorali, e il sottosegretario Castelli, che dice che utilizzeremo il bancomat o una app; ma, se qualcuno va da Unieuro, gli mandiamo la Guardia di finanza. Ma, se non hai il telefonino, come puoi utilizzare la app? Lasciamo perdere queste cose. Non parlo della pensione di cittadinanza di 780 euro, che può sembrare una cosa positiva, per invalidi civili, pensionati sociali, integrati al minimo; riguarda categorie di persone che non hanno mai versato contributi e ciò significa che andrà tutta a carico delle nuove generazioni.

questo farà sì che, per finanziarla per un milione e mezzo di autonomi, si rischia di far pagare di più a 3,2 milioni di professionisti e piccoli imprenditori. Voglio però parlare della cosiddetta pace fiscale. Va bene che rientra nei cosiddetti 12 collegati; 12 collegati non si erano mai visti e sappiamo anche che lo strumento del collegato - c'è un bell'articolo oggi su «Il Giornale» che ce lo ricorda - permette di posticipare l'entrata in vigore e gli effetti di queste Non voglio dire che il vice presidente Di Maio parla di un ragionamento di saldo e stralcio per i padri di famiglia che si trovano vessati dall'Agenzia delle entrate, mentre il vice presidente Salvini parla di un condono tombale, prima fino a 5 milioni, poi fino a un milione,

Purtroppo ha ragione sul condono fiscale tombale, ma non sui 35 miliardi. Qual è però il problema? Il problema è che l'effetto annunciato sta intaccando il gettito fiscale da contrasto all'evasione in maniera significativa, per una cifra approssimativa di quasi 4 miliardi. È aumentato automaticamente il partito del «non pago, tanto arriva il condono»; il fisco si sta congelando e si rischia di vanificare gli sforzi degli ultimi anni di lotta all'evasione fiscale. che nel 2014, certificata dal Governo, era pari a 112 miliardi, nel 2015 a 107 miliardi e nel 2017 a 91 miliardi. Ecco, con questo effetto annuncio noi stiamo non solo cancellando il lavoro passato, ma anche producendo dei danni diretti alle entrate fiscali. Coloro che hanno aderito alla rottamazione *bis* prima del 15 maggio e hanno pagato la prima rata il 31 luglio quale interesse hanno adesso a continuare a pagare le altre? Hanno l'interesse che hanno ottenuto il blocco dei pignoramenti e delle ganasce e la possibilità di ottenere il DURC; ma questo significa 600 milioni in meno di entrate. Coloro che nel maggio 2015 avevano una cartella, ma hanno deciso di non partecipare alla rottamazione, vista l'aria del condono, hanno rinunciato allo sconto del 35 per cento. I contribuenti in regola, che avevano ricevuto delle lettere e che quindi avevano iniziato un'interlocuzione

Questi sono i fatti che hanno già iniziato a danneggiare il Paese, un Paese che voi state disgregando, commettendo fondamentalmente due errori: ieri, nell'aver fatto promesse elettorali irrealizzabili, sapendo che erano tali, e oggi facendo finta di crederci per mascherare una campagna elettorale che duri fino alle elezioni europee, per trasformarle in un giudizio di Dio, in una vera e propria ordalia, dove chi rischia di non sopravvivere non siete voi, ma il Paese. E questo - guardate - l'Italia proprio non lo merita.

stiamo semplicemente parlando di una manovra a debito - tutta a debito - per spese correnti. Questo è il succo. Se mi dovessi esprimere in modo sintetico, ma comprensibile ai cittadini, è come se una famiglia già fortissimamente indebitata tornasse da tornasse da coloro che già le hanno prestato soldi - cognati, amici, sorelle - per chiederne di più, ma non

Non c'è neanche un profumo di investimento - se guardo i dati della Banca d'Italia, stiamo parlando dello 0,2 per cento - con sovrano disprezzo persino della matematica e dell'aritmetica. In più,

ma perché milioni di investitori e risparmiatori, italiani e stranieri, ritengono che il nostro debito sia diventato rischioso. È molto semplice. Lo fareste anche voi. Lo *spread* è una cosa molto concreta, non è negli arcani bancari chissà dove: è una cosa molto concreta, che riguarda tutti i cittadini e danneggia le persone più povere. Possiamo anche dichiarare che abbiamo risolto il problema della povertà, ma non è così, perché lo stiamo semplicemente alimentando. Infatti, lo *spread* aumenta il costo del debito pubblico quindi, aumenta le tasse per i cittadini: più *spread* uguale più tasse; diminuisce il valore dei titoli di Stato detenuti e dunque il valore degli investimenti: più *spread* uguale meno risparmi; aumenta il tasso di interesse sui prestiti e sui mutui e la disponibilità di credito per le imprese e le famiglie: più *spread* uguale meno credito; aumenta il costo degli investimenti per le società che gestiscono servizi pubblici, acqua, gas, energia elettrica, con aumento delle bollette: più *spread* uguale più rincari. Insomma, nessun cittadino guadagna qualcosa; quasi tutti ci perdono; alcuni, i più fragili, ci perdono moltissimo. Questo è quello che abbiamo di fronte a noi il malsano disprezzo delle cifre con millantate crescite a cui francamente non so chi faccia finta di credere perché è veramente dura, credo dia la situazione e la fotografia completa.

ci state facendo male da soli. Ricordate bene che il popolo, i 17 milioni che vi hanno votato, non è il popolo italiano complessivamente.

Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, siamo stati facili profeti nel prevedere qualche settimana fa le stroncature unanimi della manovra finanziaria che il Governo intende varare oggi in quest'Aula. La Banca d'Italia, la Corte dei conti, l'ISTAT, l'Ufficio parlamentare di bilancio hanno bocciato con convinzione i provvedimenti proposti, ritenendoli fondati su previsioni eccessivamente ottimistiche che non trovano delle basi concrete, alla luce dell'attuale congiuntura economica del nostro Paese, ma anche della congiuntura economica internazionale. Nel mio intervento mi preme sottolineare un aspetto importante, un concetto di responsabilità che oggi è del tutto assente dai programmi e direi dagli atteggiamenti di chi sembra oramai rapito da un'euforia incontenibile espressa con comportamenti che sono istituzionalmente censurabili, come i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E lo vogliamo ricordare perché questa manovra sarà ricordata per il balcone di Palazzo Chigi. discorsi e atteggiamenti irresponsabili e inaccettabili, che esasperano la peggiore declinazione del populismo tanto caro a questo Governo, poiché lasciano intendere che ogni desiderio del popolo, per ipotesi anche folle e assurdo ma legittimato da sufficiente sostegno numerico nelle urne, trovi in ciò la propria legittimazione. Dimenticano così che la nostra (per fortuna), è ancora una democrazia rappresentativa in cui tutti i cittadini delegano con il proprio voto la guida del Paese a chi ritengono saprà meglio decidere nell'interesse generale, e non di parte; non è una dittatura della maggioranza che, arrivata al potere, si preoccupa soltanto di saldare i propri debiti elettorali a discapito dell'intera collettività. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Purtroppo abbiamo già sostenuto più volte in quest'Aula che gran parte della manovra risente proprio di questa impostazione, per rivendicare la quale si è persino disposti a rischiare l'azzardo dei conti pubblici, pur di continuare a mascherare il *bluff* in cui purtroppo tanti elettori sono stati indotti a credere. Per chiarire quanto siano, non solo inutili, ma deleterie le scelte del Governo, vorrei citare soltanto un piccolo esempio numerico. Non volevo parlare di numeri oggi, ma deve essere un esempio chiaro. A marzo, prima delle elezioni, il famoso differenziale tra i BTP e *bund* era di 130 punti base, mentre negli ultimi giorni siamo arrivati a oltre 300. Ogni 100 punti di aumento dello *spread* ci costa in interessi 1,8 miliardi per quest'anno, 4,5 miliardi per il secondo anno e 6,6 miliardi per il terzo anno. Ciò vuol dire che la spesa di interessi crescerà enormemente per il nostro Paese. La famosa differenza, che voi oggi festeggiate, di aumento del debito pubblico la pagheranno cioè i cittadini italiani con gli interessi che dovranno pagare da questo differenziale; quindi, tutto quanto sarà stesso debito. Dunque, una manovra del popolo, sì, ma nel senso che sarà pagata interamente dal popolo, soprattutto da chi lavora e produce, da tutti coloro che nei prossimi mesi andranno in banca ad accendere i mutui, a chiedere un prestito che poi dovranno rimborsare con degli interessi più alti, da tutti quei contribuenti che non potranno più detrarre dai redditi le spese mediche, universitarie e gli interessi passivi. Se dovessi sintetizzare con una immagine, questa è una manovra che con una mano elargisce una mancia elettorale e con l'altra, di nascosto, sottrae il portafoglio agli italiani Ma entrando nello specifico delle nostre proposte - in quest'Aula noi facciamo opposizione costruttiva e non la facciamo, a prescindere, dal ruolo di opposizione - noi abbiamo chiesto e vogliamo oggi, con la nostra risoluzione, approvare delle proposte concrete. Noi chiediamo di adottare dei criteri di riduzione della spesa pubblica di tipo selettivo. Noi chiediamo di tutelare il risparmio degli italiani e prevedere delle forme di detassazione. Noi chiediamo di riformare il sistema tributario con la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e per le imprese e di adottare provvedimenti in grado di perseguire l'obiettivo della crescita. Noi chiediamo, soprattutto, di aumentare i posti di lavoro introducendo la detassazione e decontribuzione per sei anni delle nuove assunzioni dei giovani. Ma soprattutto, infine, noi chiediamo di attuare un grande piano strategico per il Sud, che consenta al Meridione di allinearsi finalmente a quelli che sono gli *standard* europei e nazionali, fondati sull'iniziativa e sul merito. Il piano deve realizzarsi attraverso misure che rilancino lo sviluppo infrastrutturale e industriale. Invece, siamo costretti a sentire, purtroppo, dalle parole del ministro Tria che il reddito di cittadinanza è il provvedimento per il Sud. Sono parole vergognose, che il Sud non merita assolutamente, che lo condannano al ruolo di assistito perenne e che non riconoscono, purtroppo, le enormi potenzialità che il Meridione potrebbe mettere in campo se venisse sostenuto con appositi e opportuni interventi1 I cittadini meridionali chiedono lavoro e interventi strutturali. I giovani e le famiglie rivendicano il diritto di programmare con serenità il proprio futuro nella propria terra, grazie a uno Stato che li sostiene creando le migliori condizioni affinché queste prospettive divengano realtà. Accontentare soltanto quella parte di elettorato che chiede di trovare una soluzione al disagio nelle promesse illusorie del reddito di cittadinanza è avvilente per il Sud, che lavora, produce e merita uno sviluppo dignitoso. Chiediamo al Governo di uscire dal vicolo cieco della campagna elettorale perenne; di togliersi i paraocchi della propria autoreferenzialità; di guardare con onestà intellettuale la complessità dei problemi e delle situazioni da affrontare e da risolvere; di prestare attenzione alle indicazioni degli operatori del settore e delle autorità che, unanimi, esprimono seria preoccupazione per gli effetti negativi delle scelte che si stanno per operare. Si abbandoni la logica dello scontro a favore del confronto e della sintesi, frutto di una dialettica costruttiva per il bene di tutto il Paese. Forza Italia chiede al Governo di avere rispetto della drammatica situazione del Paese, con una disoccupazione giovanile pesante che oggi è aggravata ancora maggiormente dal famoso decreto dignità. Chiede rispetto nei confronti degli italiani, che vivono giorni difficili e che hanno bisogno di soluzioni concrete e non di teatrini squallidi o di tristi feste un balcone accompagnate da surreali dichiarazioni.

la manovra del popolo nella Nota di aggiornamento al DEF presenta una spesa di 36,7 miliardi nel 2019, di cui 21,5 distribuiti con misure sacrosante, mai ideate in precedenza, pari a 9 miliardi sul reddito e pensione di cittadinanza;

un miliardo per le assunzioni nelle Forze dell'ordine e 1,5 miliardi di euro dai fondi dormienti per risarcire i truffati dalle banche dopo l'esproprio del risparmio, denominato *bail in*, che ha addossato a migliaia di famiglie gestioni fraudolente del risparmio e offerto un salvacondotto ai bancarottieri. che hanno messo in mezzo a una strada persone e hanno avuto anche una buonuscita milionaria. E ricordiamo l'immunità alle autorità vigilanti, Consob e Bankitalia. Questa è una netta inversione di tendenza rispetto alle precedenti manovre a favore dei soliti noti. In particolare dal 2013, Governi e Parlamento hanno legiferato per scardinare diritti economici e sociali, con decine di provvedimenti a favore delle banche, nel solco di una dottrina totalitaria neoliberista, introdotta negli Stati Uniti da Milton Friedman, che ha sostituito la sovranità popolare con la sovranità di mercato, la prevalenza dell'economia sul diritto e sulle Costituzioni, relegando gli uomini a merci, e ricordiamo il *jobs act* *(Applausi dal Gruppo M5S)*; una ideologia che ha corrotto la società, favorito le disuguaglianze, privatizzato i beni comuni e condotto l'economia in una delle più gravi recessioni della storia. Milioni di italiani, impoveriti da queste politiche economiche di Governi fedeli esecutori dei programmi di *troika* e cleptocrazia europea su *fiscal compact*, pareggio di bilancio, con vecchi che non si possono curare e vivono sulla propria pelle condizioni di sofferenza e grave disagio sociale,

che rappresenta - colleghi - non un regalo ai fannulloni, bensì una necessità presente in tutti i Paesi europei, perché funzionale a quella tanto decantata economia di mercato che, dopo la distruzione di posti di lavoro da parte di informatica, robotica e intelligenza artificiale, distribuisce redditi per alimentare i consumi e l'ordinato ciclo economico. Le coperture ci sono, basta leggere il DEF. Abbiamo ereditato le famose clausole di salvaguardia che facevano scattare l'aumento automatico dell'IVA a 12,5 miliardi di euro nel 2019, introdotto per la prima volta nel 2011 dal Governo Berlusconi, assieme a quel macigno del debito pubblico - 38.000 euro su ognuno dei 60 milioni di abitanti cheè stato aumentato nella scorsa legislatura di 261 miliardi, 4,3 miliardi di euro al mese

Negli Stati Uniti del populista Trump, le cui misure economiche espansive non tradizionali hanno rimesso in moto la crescita e un periodo di prosperità mai visti prima nel breve tempo del suo Governo, viene evocato il quinto emendamento per evitare che eventuali risposte possano essere usate contro i cittadini oggetti di indagini giudiziarie. A noi, signor Presidente, colleghi, piace evocare l'articolo 1 di quella Costituzione che abbiamo strenuamente difeso nel *referendum* del 4 dicembre 2016, con la Repubblica fondata sul lavoro e la sovranità che appartiene ai popoli, Gruppo M5S)*, al globalismo delle povertà, alle multinazionali, al neoliberismo dittatoriale, ai banchieri di affari, *troika*, Bankitalia, agenzie di *rating* e brigatisti della finanza criminale, che tentano di rendere inutile il suffragio universale.

noi riaffermeremo il primato della politica e dei Governi eletti su tecnocrazie e neoliberismo dittatoriale, che umiliano la dignità del lavoro di donne e uomini, per conseguire profitti sulla pelle dei popoli liberi che rifiutano di essere schiavizzati,

che stanno diffondendo a piene mani nel Paese ci porterà al disastro e all'impoverimento di quel popolo che si vorrebbe favorire. Mi concentro invece soprattutto sulla parte infrastrutturale del DEF. Intanto una certezza davanti all'Italia ed è bene che essa lo sappia: nel DEF sono previsti investimenti nei prossimi quindici anni per 150 miliardi di euro, di cui 100 immediatamente a disposizione, già presenti nelle casse dello Stato. Ebbene non c'è un euro in più da parte del Governo nel programma degli investimenti perché ciò che è inserito nel DEF non sono altro che il programma e gli interventi già previsti dal precedente Governo. Questo ci fa dire che al momento, se non per il blocco di alcune opere, sulle quali tornerò tra poco, non avete previsto alcunché per lo sviluppo del Paese, anzi, per il 2019 prevedete una riduzione degli investimenti pubblici pari allo 0,2 per cento. È bene che questo nel nostro Paese si sappia. Nel DEF vi sono però altre sciagure, come quella di mettere le mani in un certo modo sul codice degli appalti. Una cosa è coniugare la velocità con la legalità, cosa è ciò che state promettendo: una *deregulation* del codice degli appalti che potrebbe comportare il ritorno del malaffare nella pubblica amministrazione.

facendo esempi concreti che dimostrano le difficoltà oggettive delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese a fare quel tipo di attività. Mi soffermo su una delle iatture contenute nel DEF: il riesame di alcune importanti infrastrutture che sono decisive per lo sviluppo del Nord del Paese, in particolare, la Gronda autostradale di Genova, la Pedemontana lombarda, il Terzo valico e il collegamento alta capacità-alta velocità tra Brescia e Padova e la Torino-Lione. Questo riesame, peraltro già fatto in particolare per la Brescia-Padova, ha già comportato nel 2015 un risparmio di circa 500 milioni di euro. I ritardi che però determinerete a causa del riesame che state facendo metteranno in ginocchio l'economia di gran gran parte del Nord del nostro Paese. Mi soffermo in particolare, non solo sulla Brescia-Verona e, quindi, il collegamento verso la Germania e il Nord Europa attraverso il Brennero, ma sul risibile risultato che otterrete per quanto riguarda il Terzo valico e la Gronda autostradale di Genova. Coloro che definivano il crollo del ponte una favoletta stanno riuscendo nel bloccare la città di Genova e il suo sviluppo per i prossimi anni.

Questo riesame causerà non pochi danni e lo dico in particolare, per tutte le opere che ho citato, ai governatori Toti, Fontana e Zaia che in questi giorni e mesi si sono "sperticati" a dire che non era vero. È la prima volta invece che in un atto ufficiale del Governo vengono sulla carta il blocco e il riesame di queste opere. Mi rivolgo a questi tre governatori perché battano un colpo: è nelle loro Regioni che si crea gran parte del prodotto interno lordo del nostro Paese. Bloccare queste infrastrutture significa nuocere all'Italia. Potrei parlare a lungo del trasporto ferroviario, soprattutto regionale, ma concludo, Presidente, visti anche i tempi. A Toninelli, che è il Ministro, in conclusione vorrei anziché preoccuparsi dei *tunnel* che non esistono (risibile la magra figura sul *tunnel* del Brennero) dovrebbe preoccuparsi del *tunnel* certo che sta determinando con la sua pianificazione al nostro Paese. *(Applausi

Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho ascoltato poco fa il senatore Lannutti del MoVimento 5 Stelle e mi stavo chiedendo quale Paese reale frequenti perché tutti i dati ottimistici che lui vede io nel Paese reale non li vedo. non li vedo. Queste manovre che sono state, con tanta protervia, preannunciate dal Governo non depongono a favore dell'ottimismo. Lo dicono non tanto soggetti vicini ma soggetti neutri, tecnici. C'è stato il no della Banca d'Italia, il no della Corte dei conti, il no da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e voi ostinatamente andate avanti. Le spese correnti non creano crescita del prodotto interno lordo: è una regola basilare per chi studia ragioneria alle superiori. Voi

Mi domando, e lo stesso ministro Tria in sede di audizione delle Commissioni congiunte l'ha detto: sono dichiarazioni edittali? Infatti, poi, le infrastrutture e le strutture degli enti locali - come ha dichiarato - sono incapaci vuoi per una burocrazia assurda, vuoi per un sistema della giustizia amministrativa lentissimo. Sono investimenti che rimangono sulla carta e come conferma parlare di investimenti pubblici e sollecitare anche tutte le aziende di Stato ad effettuare investimenti senza una programmazione netta e chiara, secondo me denota una leggerezza di approccio davvero molto pericolosa,

il *tunnel* del Brennero, l'alta velocità Brescia-Verona, l'alta velocità Lione-Torino, tutti progetti che devono ripartire ripartire velocemente per permettere al nostro Paese il recupero di quel *gap* infrastrutturale che ci pone fra gli ultimi paesi a livello europeo.

nell'azione mediatrice del ministro Tria e del ministro Savona, gli unici Ministri che ci danno un po' di fiducia, perché portino a ordine una situazione che sembra molto disordinata, confusa e solo populista.

un sindaco di un piccolo Comune - Concamarise in provincia di Verona - un sindaco del territorio della Bassa Veronese, un semplice amministratore che, come molti altri, fra mille difficoltà, ogni energia a propria disposizione per onorare la propria comunità, guadagnandosi il titolo di tuttofare. Non sono il solo a fare questo. Ogni giorno moltissimi sindaci sono obbligati a farlo, condividendo con i propri concittadini momenti di difficoltà e gioie. Sono qui a ricoprire il ruolo di parlamentare non per fregiarmi di un titolo, non per dettare una mia linea politica o quella del partito di cui faccio parte, ma per portare in questa istituzione, nel Senato della Repubblica, la voce e le opinioni politiche della gente dei territori. Si tratta di gente in questi anni privata della speranza di un futuro migliore, della fiducia verso la classe politica; sviliteda imposizioni arrivate dall'alto, soprattutto con continui arrivi dei cosiddetti richiedenti asilo, spesso su territori attanagliati della crisi, dove l'impresa economica dell'accoglienza diventava il simbolo della Nazione che periva: un *business* economico perpetrato ai danni degli italiani in difficoltà, per di più con la beffa di sentirsi ripetere che la diminuzione del flusso migratorio avrebbe avuto l'effetto di incrementare il debito, che la futura manodopera derivante dagli sbarchi risultasse indispensabile, per una forte necessità di lavoratori giovani che paghino i contributi. Ma ora qualcosa è cambiato. Per chi i territori li vive - come noi della Lega - non passa giorno in cui, incontrando tantissime persone, non si ricevano parole di incoraggiamento, consapevoli delle continue cannonate di una certa classe politico-economica. Persone che, come loro stesse affermano, sono tornate a sperare: «Non mollate, mi raccomando, avete tutta la nostra fiducia e stima». Queste sono le loro parole: «Riferisci a Salvini di non arretrare di un centimetro. Siamo tutti con lui». *(Applausi Persone toccate nel vivo, abusate nei risparmi bancari di una vita da una scellerata classe politico-economica spietata e crudele. Noi della Lega siamo qui per mettere al centro gli italiani con questa manovra economico-finanziaria del buon senso che il Governo ha calibrato con parametri prudenziali e non ottimistici, pur non nascondendo eventuali migliori risultati. Noi della Lega siamo qui per assumercene piena responsabilità. Il tempo dirà la sua. Come pazienti agricoltori stiamo seminando, lavorando con impegno, passione, coraggio, insieme a questo Governo, grazie al quale, gli italiani che pazientemente stanno attendendo, potranno, nel prossimo futuro, raccoglierne i frutti.

mai vista una tempesta così perfetta. Ci vuole impegno, davvero tanto impegno, a incassare cinque giudizi negativi, anzi sei, forse di più: la BCE, il Fondo monetario, la Corte dei conti, Bankitalia, la Commissione europea; da ultimo, l'Ufficio parlamentare di bilancio: per Di Maio - questa è la grande novità - tutti potenziali candidati alle prossime elezioni. Sarà davvero una grande partita; un poker e sei carte questa volta perdenti, ahimè; un poker che può portare il Paese alla rovina,

Di Maio e Salvini, perché parliamo di risorse del «popolo», parola da voi abusata, parola da voi strattonata continuamente; ma il popolo è fatto di persone, di volti: sono i lavoratori, le famiglie, gli imprenditori, i giovani. Ecco, voi volete mettere le mani nelle tasche del popolo, sui loro

un quadro di valori, come la nostra Carta costituzionale, che continuate a calpestare; una visione di futuro e - devo dirvelo - il principio di realtà, che vuol dire fare i conti con le risorse che si

reddito di cittadinanza, la bandiera del MoVimento 5 Stelle, il vostro progetto si affida ai centri per l'impiego, che - ahimè - sono inadeguati a sopportare un tale carico; e così, tutto rischia di trasformarsi in una valanga incredibile di elargizioni assistenzialistiche.

Sono scomparsi i sindaci non soltanto dalle tribune nei giorni scorsi, ma anche dai vostri progetti. Son scomparsi persino i poveri, che non sono da trattare come beneficiari, ma devono essere chiamati ad essere protagonisti della loro vicenda e della loro capacità di uscire dalla povertà.

a disposizione del principe di turno, cioè voi stessi. La parola dignità, come quella di cittadinanza, a voi molto cara, meriterebbe più rispetto: noi con il reddito di inclusione (REI) avevamo introdotto uno strumento innovativo,

su quello per la non autosufficienza e su quello per il sostegno alla vita indipendente ci farete avere delle cifre, no? Su questi temi, nella precedente legislatura ci avete combattuto, dichiarando continuamente che quei fondi erano insufficienti: ebbene, ci aspettiamo che nella legge di bilancio siano rifinanziati ampiamente. Che dire delle famiglie, evocate continuamente in questi giorni? Ci farete avere dati, elenchi e numeri certi sulla maternità, sulla fiscalità agevolata, sul quoziente familiare, sul «dopo di noi», sul *caregiver* familiare? Ci farete avere qualche dato e qualche numerino,

In conclusione, su questi temi ci siamo stati per cinque anni e ci stiamo ancora. Il PD ha consegnato e depositato qui al Senato e anche alla Camera progetti di legge che entravano nel merito di questi temi. Non vi faremo sconti

che vuole avvelenare il cuore degli italiani, impedendo loro di pensare alla buona politica. Tra il vostro dire e fare e tra il vostro dire e pensare non c'è un mare, ahimè: non c'è proprio nulla!

colleghi, oggi siamo chiamati a esprimerci e stiamo discutendo e ragionando di un documento eminentemente politico, che è l'autorizzazione

eminentemente politico e necessariamente generico. Questo documento ci racconta degli intendimenti del Governo uscito rocambolescamente dalle urne riguardo al bilancio, che arriverà nei prossimi giorni e che riguarderà i conti

quindi, in questo momento ci stiamo esercitando in un legittimo processo alle intenzioni. Di questo evidentemente dobbiamo parlare. Io mi vorrei attenere all'argomento, non anticipare i ragionamenti che faremo sulla base dei numeri che ci verranno presentati tra qualche giorno

o, meglio, si anticipa che si intende aggredire uno dei due macroproblemi che attanagliano in questo momento la sanità italiana. macroproblemi, non problemi che ne compromettono il funzionamento, ma problemi che hanno al loro interno la possibilità di far collassare il sistema. Il primo dei problemi, che ahimè non è toccato è

personale. Esso propone di ridefinire i fabbisogni e l'accesso dei medici al Servizio sanitario nazionale attraverso l'approvazione di un intervento normativo entro il 2018 il 2018 - che finisce fra tre mesi - e completando i processi di assunzione e stabilizzazione aumentando le borse di studio a favore della formazione dei giovani medici. Colleghi, questo è un problema serissimo

Su questo argomento, peraltro, interviene la famosa quota 100, alla quale noi non siamo per nulla contrari. Aspettiamo di vederla declinata positivamente, ma ma qualora quota 100 andasse in porto è stato stimato che circa il 25 per cento dell'attuale personale sanitario in servizio,

credo che nel momento in cui si apre la discussione sul numero chiuso, ad esempio, e sui *test* di ingresso alla facoltà di medicina si fa un'operazione seria; seria; decliniamola positivamente nei prossimi giorni per capire come allargare il numero chiuso.

prima esageriamo su un lato e poi sull'altro. Il numero chiuso va riprogrammato; vanno riaccordate risorse importanti alle università; vanno ripristinate le strutture per formare più medici;

nel problema. Riformare il sistema del numero chiuso significa anche rivedere tutta la vicenda dei test d'ingresso. Su questo noi aspettiamo di leggere il disegno di legge di bilancio che la maggioranza ci presenterà entro il 20 ottobre.

Un secondo argomento molto interessante che viene aperto con questo documento riguarda il tavolo tecnico di lavoro su farmaci e dispositivi medici avente in via prioritaria il compito di individuare adeguate soluzioni e modalità di ricalcolo del *payback*. Colleghi, non sono quanti di voi si occupano di sanità, ma vi garantisco che

costituirebbero un importante passo in avanti dell'attività legislativa che accompagna questi documenti. Ciò non potrebbe non indurci ad assumere un diverso atteggiamento nei confronti del Documento di economia e finanza che in questo momento evidentemente - ma lo dirà molto meglio di me il collega Marsilio, che interverrà in dichiarazioni di voto - non può che essere negativo e di censura, anche perché

in modo preoccupante tutti gli sprazzi di luce che, invece, vengono delineati dai colleghi della maggioranza. *(Applausi

ma non credo a come è stato presentato, lavorato e reso inutilmente resistente a tutte le critiche che sono intervenute.

per la condotta che si è tenuta in Commissione, ma vedo adesso anche il disinteresse in Aula, così come ho visto anche il disinteresse rispetto alle censure di organismi terzi imparziali, internazionali e nazionali. Noi sappiamo che la Nota di aggiornamento del DEF non è la liturgia di una tipografia dello Stato. La Nota di aggiornamento al DEF dà luogo ad analisi e prefigurazioni, stabilisce obiettivi e organizza la legislazione successiva.

(che secondo me assomiglia quasi ad un giubileo fiscale) della pacificazione fiscale. Adesso proviamo a dare numeri, nomi e cognomi a ciò cui può

entrate tributarie per 505 miliardi di euro e al lordo dei contributi sociali siamo arrivati a 816 miliardi di euro, mentre sono pari a 10 miliardi di euro i risultati della lotta all'evasione. Quale sarà il risultato della pacificazione fiscale? Darà luogo a gonfiezza il primo anno e inconsistenza, impoverimento di entrate negli anni successivi, oltre al carico di diseducazione, di caduta verticale di quella moralità che caratterizza il patto tra cittadini e ordinamento per quanto riguarda la coppia diritti-doveri. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Si fa una grande scommessa sul rilancio degli investimenti. In quest'Aula c'è una parte caratterizzata da esperienze amministrative e decisionali precedenti e c'è una parte che è arrivata dalla

che io ho letto sia nella stesura del MEF (che consente di scaricare il documento di aggiornamento) e anche nella parte che è stata redatta

a sostenere che, per quanto riguarda il rilancio degli investimenti, accanto alle responsabilità burocratiche, verrà prevista ed insediata una autorità di *leadership* politica che si fa carico di pianificare, programmare e gestire gli investimenti? È la caduta verticale del diritto! Si rinuncia all'ordinamento, si dà luogo ad una intromissione della politica nelle procedure. Se avessi letto da giornalista, studioso e studente all'esterno e non avessi seguito quello che accaduto qui quanto al danno circa il bando periferie, non avrei creduto possibile leggere, capire e dare luogo a quel significato. In Italia c'è una distinzione tra ordinamento e politica, statualità e politica: le procedure sono dello Stato, la maggioranza è della politica: non è immaginabile che la politica si intrometta. Non è possibile che le procedure vengano azzerate e si dia luogo ad un nuovo inizio da capo! Ma quali investimenti possono ripartire con questa cultura dell'assalto? Peraltro, l'assalto alle procedure lo avete fatto su 1,6 miliardi di euro riguardanti le città e 20 milioni di cittadini. Il moltiplicatore per le opere pubbliche è cinque; avremmo avuto una ricaduta fatta di occupazione, di sentimento positivo, di pervasività economica; invece avete voluto un azzeramento. Su questo e per questo vi dico fermatevi, rileggete, studiate, approfondite, confrontatevi, siate onesti culturalmente. Questo documento non è una recita, una liturgia, un'opera di abbellimento documentale; è un pezzo della procedura sul bilancio e del bilancio dello Stato. Per questo io dico di darci da fare con maggiore "curvatura" delle nostre intelligenze. In Commissione è stato proprio un appalto dell'inutile. Evitiamo che qui ci sia l'appalto dell'inutile! Diamoci da fare!

o forse no, nel senso che nel documento politico che è stato prodotto di programmazione intesa come volontà di riforma del sistema economico finanziario *in melius* non c'è nulla: propaganda, *slogan*, eccesso di assistenzialismo, tanti soldi spesi male: 37 miliardi, di cui 22 sono in *deficit*. Partiamo dal reddito di cittadinanza, che si è realizzato, come pare evidente, in forma di pura misura di assistenzialismo a pioggia, anzi a pioggerellina, quella pioggerellina inutile che non fa crescere nulla. Esso si trasforma così in uno strumento pericolosissimo per un Paese che ha una crisi lavorativa e produttiva profonda e perdurante; strumento che manderà in crisi, tra l'altro, il reale sistema del *welfare*. Questo sistema non aiuterà certo la ripresa, favorendo la diffusione di una mentalità passiva, perché un popolo che riceve soldi senza produrre e senza sentire la necessità di essere attivo produce solo debito. Chi di noi non vorrebbe abolire la povertà nel Paese? Ma non in questo modo, non stanziando tanti soldi che saranno tolti a tanti settori importanti per la crescita reale e la produttività. Per dare poco ai singoli, si toglierà tanto ai servizi per il Paese. Questo progetto di manovra non ci piace, perché crea false illusioni; e questo non va bene. *(Applausi dal afferma che abolirà la povertà, egli illude le persone, che dall'illusione passeranno presto alla delusione. E questo è male, perché, così facendo gli ultimi rimarranno ultimi e, nonostante l'uso di tanti soldi, il reddito di cittadinanza si trasformerà in debito di cittadinanza. Le imprese Le imprese si troveranno sempre più in difficoltà e chiuderanno o se ne andranno altrove, mentre i posti di lavoro saranno sempre meno, come sta succedendo oggi per l'*impasse* decisionale del Ministro dell'ambiente, inneggia al sostegno all'economia circolare, ma non emana alcun decreto per sbloccare le autorizzazioni *end of waste* per il riciclo dei rifiuti, che giacciono stoccati presso gli impianti fermi, con molti soggetti che stanno gridando per avere aiuto, da Legambiente a Confindustria, passando per le associazioni. E intanto si perdono soldi e posti di lavoro. Il documento del Governo in tema ambientale non contiene una sola parola sulla drammatica situazione della qualità dell'aria nella Pianura padana e nelle Regioni del Nord in generale; forse è inserita nella voce «infrazioni comunitarie», ma comunque è una grave carenza, considerando i costi sanitari e sociali che comporta. Difficile è poi parlare bene di questa *flat tax*. Amici della Lega, voi avete firmato con noi e con Fratelli d'Italia un programma che prevedeva una vera *flat tax* e non questa specie di operazione che da un lato dà e dall'altro toglie per dieci volte. Non basta chiamare le cose semplicemente con un nome perché si realizzino gli intenti; una vera e necessaria riforma fiscale non c'è e manca una vera riforma strutturale: c'è solo un leggero ritocchino, che riguarda pochi. A quale pagina, ad esempio, si legge del taglio e della riforma delle accise, tanto sbandierato? Io non lo trovo; magari potete aiutarmi voi. Ma intanto il costo dei carburanti aumenta e pesa sul bilancio familiare e delle imprese. Credo che i 5 Stelle abbiano cannibalizzato questo provvedimento e spero che il resto del Governo se ne renda conto. Abbiamo sempre dichiarato che avremmo votato provvedimento per provvedimento, ma, dopo il decreto dignità, che ha solo iniziato a mettere in crisi il mondo del lavoro, ora tocca a questa manovra terminare l'opera. Noi non possiamo che cercare di dare il nostro contributo, rendendoci conto del fatto che tutti i punti condivisi all'interno del programma di centro-destra sono stati depotenziati e sacrificati sull'altare del programma della parte gialla. Pace fiscale e pace burocratica passano attraverso la libertà del singolo, attraverso il rispetto del cittadino e non attraverso una debordante iniziativa parlamentare come quella dei 5 Stelle, che per ogni cosa pensano a una legge, andando in senso preciso e contrario a qualsiasi logica liberale e cercando di arrivare a uno Stato etico oppressivo e invasivo, che regola ogni aspetto della vita dei cittadini. Le critiche sono sempre facili. Le proposte e le soluzioni per noi non stanno nell'utilizzo incosciente della spesa corrente, ma nell'investimento per far diminuire il costo del lavoro, per ridurre il cuneo fiscale e il costo dell'energia, per aiutare le imprese, che sono il bacino dei posti di lavoro. Questo DEF comunque un cambiamento lo ha già prodotto: ha già prodotto debiti e l'erosione dei pochi risparmi degli italiani. Siete ancora in tempo. Ascoltate i nostri suggerimenti e non chiudetevi a riccio: c'è una Nazione da salvare.

signori del Governo, noi che tifiamo Italia e tifiamo per gli italiani vi vogliamo dire con molta determinazione che la vostra manovra è pericolosa. È pericolosa non solo perché è a debito, ma perché manca di un impianto strategico. Mancano misure per stimolare la crescita economica e sostenere quelle imprese che innovano, scommettono sul futuro, creano opportunità di lavoro, internazionalizzano e vanno a conquistare nuovi mercati. Mancano misure per ridurre il divario territoriale. Signor Presidente, pretendo di essere ascoltata dal

avete cancellato il Mezzogiorno. Una sola volta la parola «Mezzogiorno» è menzionata nel vostro provvedimento. Di Maio, per giustificare questa disattenzione, ha fatto una battuta a effetto: il Sud non è una riserva indiana. Certo, proprio perché il Sud non è una riserva indiana, servono interventi seri e in continuità, se non avete idee nuove. Almeno avreste potuto utilizzare quel patrimonio di idee e strumentazione che vi è stato lasciato

per la ricerca e lo sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese, che da sole non ce la fanno. Potevate rafforzare il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi macchinari,

Dovevate mantenere fede a un impegno solenne assunto dal vostro Ministro per il Sud sulla decontribuzione al 100 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Non vi è traccia di questo provvedimento. Vi do un consiglio: non invitate il Ministro solo alle feste dal balcone, ricordatevi di invitarla anche alle sedute del Consiglio dei ministri. Potevate fare un intervento, così come vi abbiamo suggerito, per tagliare il costo del lavoro a tempo indeterminato, mentre avete solo aumentato il costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato. Bisognava e bisogna fare interventi seri per innovare la manifattura, i servizi di qualità e l'agricoltura, perché l'emergenza che questo Paese ha si chiama lavoro

Di Maio, che ha una diffidenza feroce verso i potenziali beneficiari, ha parlato di sei anni di carcere. Ascoltate, cittadini e cittadine, che li avete votati: condono per i ricchi e per gli evasori, carcere per i poveri non revoca del finanziamento, ma carcere. Si potrebbero sprecare le battute, ma io invece vi voglio fare una domanda: non vi vergognate neanche un po' di questa deriva sulla quale vi siete collocati?

Avete allora conquistato meritatamente un titolo: non quello di innovatori, non di Governo del cambiamento, ma di ladri del futuro.

per me è sempre un'emozione e un privilegio prendere la parola in quest'Aula, per quello che il Parlamento rappresenta nelle nostre istituzioni democratiche, ma oggi l'emozione è doppia perché fra poche ore si compirà il primo passo di un lungo cammino verso il piccolo, grande sogno che aveva un gruppo di donne e di uomini che poi avrebbe costituito il MoVimento 5 Stelle: il sogno di far riavvicinare i cittadini alla politica, quella con la «P» maiuscola, quella che rimette al centro delle azioni e delle istituzioni le persone e le loro necessità. Un'attività nobile e semplice allo stesso tempo, che ha l'unico scopo di far vivere meglio le donne e gli uomini, e per far questo deve considerarli come individui sovrani nel loro complesso e non come sudditi da vessare. Oggi siamo alla prima vera tappa di questo cammino e abbiamo l'occasione di tramutare in realtà alcune delle idee e dei sogni del MoVimento 5 Stelle: il sogno di migliorare la qualità della vita di tanti italiani, di mantenere fede agli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Le misure della NADEF sono state ben illustrate dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto, da ultimo dal collega Lannutti, quindi non le ripeterò. Noi siamo convinti che il complesso di queste misure risponda a criteri di giustizia sociale e di equità, e porterà il Paese ad una crescita più forte e duratura. come ha affermato in audizione il vice direttore della Banca d'Italia, una crescita più sostenuta e una maggiore coesione sociale non sono in contrasto con la disciplina di bilancio:

o dare il reddito di cittadinanza a chi è in condizioni di povertà, nonché la possibilità che circolino più soldi nell'economia reale, rendono più semplice e più veloce il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati europei, che prevedono per esempio un rapporto *deficit*-PIL che non debba superare il 3 per cento, e un rapporto debito-PIL che debba tendere al 60

il Paese alla rovina esponendolo alla speculazione internazionale; che sarà difficile rifinanziare il debito pubblico perché saremo meno credibili per i mercati; che in buona sostanza siamo degli irresponsabili e stiamo regalando soldi ai poveri, e secondo loro non ce lo possiamo permettere in questo momento e in questa misura; che stiamo interrompendo - udite, udite - il ciclo virtuoso messo in campo dai precedenti Governi. Mi domando: questi punti di vista, che sono ovviamente rispettabili ma che noi non condividiamo, sono corroborati da riscontri fattuali e dai numeri, oppure sono degli esercizi di fallaci teorie economiche? Le politiche di austerità che sono state imposte al nostro Paese dal 2011 e il conseguente, significativo aumento della povertà, il tragico peggioramento delle condizioni di vita di tanti italiani hanno portato - almeno questo - beneficio nei conti pubblici? No, assolutamente no. E lo dimostrano i numeri degli ultimi dieci anni, in particolare proprio quello del rapporto debito-PIL, che - lo ricordo ancora - per i Trattati deve diminuire significativamente e tendere al valore del 60

E, infatti, nel 2010, invece di scendere, è salito ancora al 115,4 per cento. Nel 2011, nonostante arrivi il professore e senatore a vita Monti, sale ancora al 116,5 per cento. Ci dissero, però, di stare tranquilli, che non era colpa dei bocconiani e del professor Monti ma del precedente Governo e che, quindi, tutti i sacrifici e l'austerità che ci imponeva l'Unione europea ci avrebbero, non solo salvato a breve, ma, anzi, ci avrebbero regalato ricchezza di lì a poco. Infatti, l'anno dopo, l'anno del Governo pieno dei bocconiani e dei professori (mica come il governo dei barbari leghisti e grillini di oggi) porta quel rapporto al 123,4.

nel 2014, anno dei Governi Letta e Renzi, si issa al 131,8, che è il massimo storico nel periodo considerato.

Ovviamente, è una situazione che noi non potevamo sopportare. Avevamo preso un impegno con i nostri elettori. Abbiamo messo in campo una manovra espansiva e siamo certi che i mercati la apprezzeranno nel brevissimo periodo. Concludo dicendo che io sono orgoglioso e felice di aver avuto il privilegio di partecipare alla formazione e all'approvazione di questa Nota di aggiornamento al DEF che, per le misure di cui traccia il quadro programmatico, costituisce la speranza di una vita migliore per milioni di nostri connazionali, che è il principale obiettivo di questa forza politica. Quando, fra qualche ora, noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle premeremo il pulsante verde, con noi lo premeranno, idealmente, i milioni di cittadini che ci hanno sostenuto e che credono in noi. E aggiungo che, insieme a noi, voteranno, anch' essi idealmente, i fondatori del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che ci guarda di lassù.

provo a fare tre considerazioni in questi pochi minuti. La prima è sulla comunicazione. Notavo, infatti, che le cose sbagliate godono del privilegio di essere spesso raccontate con parole semplici, mentre le cose giuste spesso non godono di questo privilegio e hanno necessità di ragionamenti frequentemente complessi. Penso, per esempio,

fisico e astronomico. Provo a spiegarlo così: anche il cartello di limite di velocità prima di una curva non è tassativo o drastico. Dice semplicemente una cosa: superare quel limite espone a dei rischi maggiori di uscire di strada. Poi, dipende dalle condizioni dell'auto che si sta guidando. Chi ha l'auto con il bagagliaio pieno di debiti corre meno rischi di chi i debiti li ha in un rimorchio carico attaccato al gancio di traino. Tutto qui. Ignorare i numerini, cioè i limiti di velocità, significa correre molti rischi di uscire di strada. Poi c'è anche da considerare chi c'è al volante. Beh, al volante ci siete voi, della Lega e del MoVimento 5 Stelle, e state facendo la manovra sbagliata, che porta il Paese nel fosso. Noi che cosa avevamo fatto Niente. COLLINA *(PD)*. Avevamo camminato su quel crinale, che peraltro è sempre quello sul quale ci troviamo ancora oggi, che ha da una parte il burrone dell'aumento del debito pubblico e dall'altra il burrone della mancanza di crescita economica. Ed è stato un esercizio di equilibrio riuscito, perché abbiamo restituito, dopo cinque anni di Governo, un Paese saldamente avviato sulla strada della diminuzione del debito e altrettanto situato in un evidente percorso di crescita economica attraverso gli investimenti sulle infrastrutture e sul territorio. Vede, senatore Lannutti, lei ha detto che abbiamo portato il Paese alla recessione, ma non è vero e il vostro voto sul consuntivo di qualche giorno fa lo certifica. Se oggi potete giocare d'azzardo con i conti del Paese dandogli una parvenza di sostenibilità, è grazie al lavoro di questi nostri Governi. Infine, un aspetto non meno importante che solo ieri abbiamo sentito, in ossequio a quanto dicevo prima, banalizzare con parole semplici. L'articolo 81 della Costituzione prevede che lo Stato assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico e che il ricorso all'indebitamento sia consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico. Su questo punto specifico, la Nota di aggiornamento è preoccupante perché teorizza una doppia violazione dell'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 81 afferma

terremoti o altro, che invece abbiamo affrontato noi nei cinque anni precedenti. Noi affermiamo, quindi, che questo DEF viola i limiti posti dalla Costituzione all'articolo 81. Bene, di fronte a questo voi andate avanti, rinunciate ad affrontare tutti gli elementi di complessità che oggi il quadro internazionale pone pone ed esponente il Paese a dei gravissimi rischi. Noi ci opporremo a questo anche con delle proposte nella prossima discussione della legge di bilancio.

la Nota di aggiornamento al DEF fa acqua da tutte le parti e sono tanti i passaggi che ci lasciano perplessi. Uno di questi è sicuramente quello che riguarda le caratteristiche che dovrebbero avere le proposte di lavoro da fare a chi percepisce il reddito di cittadinanza, strumento che tra l'altro consideriamo meramente assistenzialista e che Forza Italia boccia *in toto.* Ebbene, nero su bianco è scritto nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che le proposte di lavoro dovranno essere eque e vorrei tanto capire cosa si intende per eque, perché è un termine molto vago che lascia spazio all'interpretazione: vuol dire tutto, ma non vuol dire nulla e poi chi stabilirà quando una proposta è equa e quando non lo è? lo è? Sempre nella Nota di aggiornamento, c'è scritto che queste proposte di lavoro non dovranno essere lontane dal luogo di residenza del potenziale lavoratore, quindi chi non accetterà una proposta di lavoro perché non sufficientemente comoda, perché non sotto casa, continuerà a percepire il reddito di cittadinanza a tempo indeterminato? Ecco, su questo punto credo che si dovrebbe fare assolutamente chiarezza, perché se questo è il messaggio che volete mandare, è un messaggio fortemente antieducativo da dare alle nuove generazioni. Anziché dire ai ragazzi che il lavoro dà dignità, quindi bisogna lavorare, rimboccarsi le maniche anche a costo di fare dei sacrifici, darsi da fare anche a costo di cambiare città, con il reddito di cittadinanza formulato in questo modo voi vi state prendendo la responsabilità di dire a questi stessi ragazzi di non accettare di lavorare se non fa loro comodo, tanto lo Stato li mantiene. Per non parlare del fatto che queste proposte di lavoro dovrebbero provenire dai centri per l'impiego, che al momento non sono messi in rete tra loro, non hanno sufficienti dotazioni informatiche e occupano solo il 3 per cento di chi vi si rivolge. Il reddito di cittadinanza, dunque, secondo i vostri calcoli, verrà distribuito subito, ma nel frattempo attenderemo che i centri per l'impiego funzionino davvero, siano efficienti e possano dare risposte concrete in termini di proposte di lavoro. Passeranno anni e il corto circuito sarà inevitabile. Voglio sottolineare che per noi di Forza Italia la lotta alla povertà è sacrosanta, ma non se fatta con questi strumenti. Se non si crea lavoro con investimenti, che nella NADEF non sono pervenuti,

partite dall'idea sbagliata che il lavoro di un giovane sia strettamente collegato alla pensione di un anziano. Partite quindi dal presupposto che il numero dei posti di lavoro sia fisso e contingentato; una contraddizione in termini, visto che vi definite il Governo del cambiamento e sostenete che le vostre ricette economiche aiuteranno la crescita del Paese.

Ci sono stati numerosi chiarimenti da parte del Governo. Credo che su questo piano sia stata chiarita l'attendibilità dei numeri proposti nel DEF. non si possano ritenere affidabili le stime del MEF oggi, con questo Governo, quando si è ritenuto sempre che lo fossero con i Governi precedenti. Lo sono oggi, come lo erano in passato. Tuttavia, al di là dei numeri, dobbiamo considerare la situazione in cui vive il Paese. La situazione economica, il benessere dei suoi cittadini e, da lì, partire per fare le scelte. è allora la situazione che fotografiamo oggi, dopo sei anni di Governi di centro-sinistra, del Partito Democratico, dei vari Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni? È la fotografia di un Paese in gravissima difficoltà. difficoltà. Si parla di crescita; la crescita non c'è, non c'è ancora. Ricordiamo che negli anni passati la crescita dell'Italia è stata un fanalino di coda a livello europeo. Voi avete avuto grandi opportunità in questa fase di poter far crescere l'economia in una situazione apparentemente più favorevole che in passato. Ma non avete agganciato la ripresa, non avete approfittato di una situazione che poteva dare delle opportunità. opportunità. Si può inoltre dire che dopo questi sei anni il livello di tassazione a carico delle imprese e delle famiglie sia diminuito? Io credo proprio di no e anche da questo punto di vista è necessario cambiare, continuare rispetto alle politiche che avete attuato negli anni passati. Rispetto poi alla disoccupazione il nostro Paese vive una situazione drammatica soprattutto a livello di giovani. Un dato che voi non citate ed ignorate costantemente è quello dell'emigrazione dei nostri cittadini; 100.000 italiani all'anno emigrano in altri Paesi in cerca di fortuna. Questo è un dato inaccettabile. Emigrano soprattutto i giovani laureati, che dovrebbero essere la speranza del nostro futuro. Il sistema pensionistico è passato da quello dell'Italia degli anni Ottanta, delle *baby* pensioni, a quello del PD degli anni 2000, che è il più alto a livello europeo. È una situazione inaccettabile che costringe

Quindi questo deve cambiare e ciò deve avvenire anche per dare l'opportunità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro ed alle imprese di avere forze nuove dotate di conoscenze legate alle necessità di questa fase storica della nostra economia. Poi c'è un altro tema che la sinistra - che voi teoricamente dovreste rappresentare - non ha affrontato ed è quello delle diseguaglianze sociali che sotto i vostri Governi sono aumentate in modo indecoroso e inaccettabile. Il divario tra ricchi e poveri è aumentato, il ceto medio non esiste più e questo grazie alle vostre politiche inesistenti da questo punto di vista. Avete strozzato gli enti locali non dando più risorse con regole assolutamente inaccettabili negli investimenti di opere pubbliche. Questo Governo ha già avviato riforme che permettono di utilizzare l'avanzo di bilancio e lo farà anche nei prossimi anni, con questo DEF e con la legge di bilancio, finalmente promuovendo investimenti. Poi c'è stata la crisi del sistema bancario, una crisi che voi avete gestito in modo irresponsabile. Con un decreto-legge, nel giro di una notte, avete cancellato i risparmi di decine di migliaia di risparmiatori. Non siete riusciti a salvare, poi successivamente, le banche venete, di fatto bruciando il frutto del lavoro di tante famiglie italiane che hanno risparmiato e che voi non avete tutelato, anzi, le avete condannate ad una situazione di povertà e di miseria. Poi c'è la politica sull'immigrazione che è stata semplicemente folle e irresponsabile. Avete trasformato l'Italia nel centro profughi d'Europa,

dal Gruppo PD)*. Questo è il dato di fatto che non è una valutazione della Lega, è una valutazione dei cittadini italiani che voi dovreste rispettare e non considerare ignoranti perché fanno scelte diverse da quelle che voi vi aspettate da loro. È un processo difficile, è un processo che richiede impegno, ma noi lo porteremo avanti con determinazione. Possiamo accettare tutto, possiamo accettare critiche da tutti, soprattutto dai cittadini che incontriamo costantemente, ma le prediche da parte vostra non le accetteremo mai. Non da chi negli ultimi sei anni ha tolto ai cittadini italiani tutte le certezze che avevano. Hanno perso ogni certezza nel futuro. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Questa è la vera sfiducia che c'è nel nostro Paese e la responsabilità è chiara.

Avete tolto loro la sicurezza di vedere al sicuro i loro risparmi, con la crisi del sistema bancario e con le scelte di cancellare i risparmi dei cittadini italiani. Avete tolto loro la certezza di una pensione che desse dignità alla loro vecchiaia, avete tolto loro la certezza di avere un lavoro dignitoso e di avere un reddito decoroso. Questa è l'incertezza che esiste nel nostro Paese. Questo è il clima di insicurezza dei nostri cittadini: un'insicurezza che deriva dalle vostre politiche, dalle politiche di Monti, le politiche delle tasse, della riforma Fornero, dei tagli agli enti locali, ma anche dei Governi successivi. Colleghi, in relazione al rapporto *deficit-*PIL voi avete attuato leggi finanziarie con *deficit* al 3 per cento, al 2,6, al 2,5, con un Renzi che teorizzava il 2,9, e solo la finanziaria di questo Governo al 2,4 dovrebbe terrorizzare i mercati, dovrebbe essere la causa di tutte le crisi del nostro Paese. *(Commenti dal Gruppo PD).* Non accettiamo questo tipo di lezione. L'Europa è un'entità che ha una Commissione

fondamentale che è stato toccato concerne la fiducia e la credibilità: anche per noi sono valori importanti. È importante la fiducia dei mercati; può esserlo, forse, quella della Commissione europea; lo è sicuramente di più quella del popolo italiano, e voi l'avete persa. Noi l'abbiamo conquistata ed è nostro dovere fare scelte coraggiose, assumerci le nostre responsabilità e governare nell'interesse Questo è il nostro unico obiettivo e governeremo solo a queste condizioni.

Signor Presidente, non c'è dubbio che la presente Nota di aggiornamento rappresenti il primo atto politico importante di questo Governo e delle maggioranza che lo sostiene. dunque, surreale, assurdo, che chi ha responsabilità di Governo continui a guardare a un'opposizione al passato, senza alcuna condizione per indicare una strada per il nostro futuro e per il futuro di questo Paese. Si continua imperterriti a confondere le responsabilità importanti che sono all'interno di questa Assemblea; si continua, cioè, a guardare alle elezioni e a trascurare le generazioni. Trovo che questo sia inaccettabile, irresponsabile, dannoso per gli italiani prima di tutto. La presente Nota di aggiornamento cambia radicalmente la strada delle politiche economiche, finanziarie, strutturali, del bilancio delle Stato. Fa un'inversione che consideriamo pericolosa, perché abbandona una strada, quella che era stata nelle condizioni - pur di fronte a un quadro macroeconomico difficile - di coniugare un sostegno alla crescita con una tenuta, un consolidamento dei conti pubblici. Colleghi, i numeri restano; le chiacchiere spariscono. Dal 2008 al 2013 abbiamo perso 9,4 punti del PIL; dal 2014 al 2017 ne abbiamo recuperati 3,7: sono sono elementi strutturali che non possono essere cancellati dalla propaganda. Qui si compie un'inversione pericolosa, insidiosa. Si spinge l'Italia, per la prima volta, in un quadro macroeconomico di cui questo provvedimento non tiene conto, completamente estraneo dal quadro macroeconomico che sta sopra di noi. cioè, l'Italia su un ottovolante, mettendo a rischio la stabilità, la credibilità e la fiducia. Per di più, all'interno di quest'Assemblea, assistiamo anche a una strumentale, insostenibile contrapposizione tra il popolo e il mercato, tra la società e l'economia, tra il pubblico e il privato; un'apertura di un conflitto innaturale, privo dei valori di riferimento, perché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, per contrastare la povertà, la strada maestra resta il sostegno al lavoro, alla crescita, allo sviluppo. contrario, questa è una manovra che configura un perimetro totalmente orientato a forme di sussidi, di assistenza, negando il futuro e contrapponendo il popolo al mercato, quando sappiamo bene che per migliorare le condizioni di vita dei cittadini occorre vivere all'interno di una comunità; occorre garantire lavoro, e il lavoro lo si garantisce attraverso gli investimenti. E dunque contrapporre il popolo al mercato è una follia e un errore grave,

con le quali si sovrastima la crescita. Altra questione fondamentale, che ci preoccupa molto, è che i moltiplicatori che avete messo a fianco del reddito di cittadinanza - e, ancor più, degli investimenti - sono irreali: irreali: i 12 collegati che avete previsto occuperanno quasi tutta la prima metà del 2019, dunque avete costruito anche previsioni insostenibili

di quest'assurda follia di chi vuole piegare l'Italia verso un qualcosa di individuale e insostenibile nelle forme assistenziali si scaricherà sulle famiglie e sulle imprese, perché si ridurrà la propensione agli investimenti all'interno della famiglia e diventerà più difficile l'accesso al credito, indispensabile per generare lavoro e crescita. Tutto questo, allora, mi porta a pensare che quando diciamo che manca una visione di futuro è perché purtroppo a pagare tale prezzo saranno i giovani, se non si cambiano orientamento e strada.

Molti di quelli che vi hanno votato forse pensavano che, visto che vi siete presentati come tali, aveste a cuore proprio il loro futuro. In realtà, dei futuristi - e quindi della visione del futuro - avete solamente le parole in libertà:

quotidianamente con i vostri monologhi via *social* possiamo contrapporre la ragione, forse un po' fredda, dei numeri.

che volete coniugare tutto all'indicativo futuro, ma che poi, con i vostri «faremo», «diremo» e «prometteremo», non realizzate niente, tre cose certe le avete già dette, grazie ai numeri che avete presentato all'interno della Nota di aggiornamento al DEF: in primo luogo, ci sono zero investimenti nel sapere, il che significa zero investimenti in cultura, università, ricerca e scuola; in secondo dal Gruppo L-SP-PSd'Az):* per ora, l'unico gesto che avete fatto è stato quello di disincentivarlo e sapete benissimo quali sono già i primi esiti del "decreto disoccupazione".

Colleghi del MoVimento 5 Stelle, avevate o no detto che avreste investito nella scuola 15 miliardi? Dov'è quella tabella? Siete in ritardo sulla tabella di marcia o c'è qualcosa che non torna? *(Applausi dal Gruppo PD)*. La scuola per ora la utilizzate solo come un bancomat

avete tagliato sulle ore di alternanza scuola-lavoro. Avete tagliato i fondi! Potevate tagliare le ore - saremmo stati contrari comunque - ma perché avete tagliato i fondi sull'alternanza scuola-lavoro? Poi ci venite a dire che per una persona che manderete in pensione un'altra la assumerete? Le aziende vogliono le competenze, che si acquisiscono attraverso l'alternanza scuola-lavoro, primo strumento per l'acquisizione delle competenze trasversali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non fate altro che disinvestire anche su Industria 4.0 e su Impresa 4.0, perché, in fondo, per voi il ricordo solo quello del passato. Scommettete su ciò che vi dà il consenso perché il cambiamento vi fa paura. Avete detto che avreste organizzato il «*team* mani di forbice». Avete iniziato dalla scuola e, quindi, vi crediamo.

I brutti e i cattivi del Partito Democratico hanno messo 14 miliardi sulla scuola. Noi non accettiamo più lezioni da nessuno e, tantomeno, da voi, che siete - ve la leggo perché la citazione chiaramente non è mia - «l'esempio più fulgido di come i rivoluzionari più radicali diventano conservatori il giorno dopo la rivoluzione».

Signor Presidente, le debbo confessare che avrei voluto fare un intervento parlando di numeri, cercando di analizzare approfonditamente alcuni aspetti salienti di questa Nota di

cui mai avrei pensato di assistere - di un Ministro dell'economia che viene silenziato dal Presidente della Commissione in piena audizione solenne: non mi sarei mai immaginato di vedere in questo Paese un Ministro dell'economia che viene allontanato dalla addetta stampa di un Ministro dell'interno per evitare un confronto con i giornalisti. Dinanzi a tutto ciò è difficile mantenere contegno e serietà.

invece, un'altra forza politica che ritiene che al centro non ci debba essere la persona, bensì lo Stato, che interviene in tutte le dinamiche economiche. Diventa assai difficile. Lo dico a scanso di equivoci: sul reddito di cittadinanza, come si fa a poter dire di no a prescindere? Ci sono sacche del Sud e tante parti del Paese che vivono grandi difficoltà e, allora, è ovvio che anche noi volevamo dare una mano. Su questo non c'è dubbio.

lo Stato. Pochi giorni fa il «Corriere della Sera» ci ha mostrato in modo drammatico che per aprire una parruccheria in Italia nel 2018 ci vogliono ancora 48 nullaosta. Voi pensate che con queste dinamiche si possano rilanciare l'economia e il PIL?

caricate il *deficit* per mantenere le promesse e avete fatto una frittata pazza, mettendo insieme un po' di *flat tax*, un po' di Fornero e un po' di reddito di cittadinanza. Questo non porterà alcun beneficio,

fa allora, Presidente, ad essere seri dinanzi ad un ministro come Toninelli, non tanto per il tunnel del Brennero, quanto per le menzogne che ha detto ai cittadini di Genova, visto che dopo

mandateci Rocco Casalino, che voi e solo voi potevate rendere il genio della comunicazione in questo Paese. quando la mattina in Commissione bilancio si presenta il vice ministro Castelli, nutro per lei un sentimento di tenerezza, vedendola devastata alle 9 del mattino,

avete attaccato i funzionari pubblici solo perché sono fedeli alla Costituzione; avete deriso professori di economia; avete persino isolato la Ragioneria generale dello Stato. A noi mortali, a noi cittadini italiani non rimane dunque che affidarci alla fortuna,

L'auspicio che noi rivolgiamo a voi, ma soprattutto ai nostri concittadini, è che quella casella rimanga un'opzione del gioco e non diventi, a causa della vostra arroganza, il destino di un'intera Nazione. Questo è il gioco che vi vogliamo regalare,

la manovra economica e la Nota di aggiornamento che la precede sono sicuramente l'impegno più gravoso di ogni Governo ed una sorta di carta d'identità. Mi lasci dire subito, signor Presidente, che i primi passi di questo Governo nella sessione più importante, che è quella di bilancio, non ci sembrano così brillanti; anzi, quello che emerge è un dato di approssimazione, di superficialità dire) persino di sciatteria. Infatti, può anche non piacerci questo modello nel quale viviamo (a noi non piace e anzi vorremmo superarlo), ma non essere consapevoli del fatto che la dichiarazione dell'ultimo dei Sottosegretari crea al Paese inutili incertezze e fibrillazione è una responsabilità che fa sì che questo Governo si dimostri non all'altezza della prova. Lo dico persino al netto del contenuto di cui ci vogliamo occupare. A mio avviso i dieci anni che sono alle nostre spalle hanno cambiato il volto di questo Paese hanno cambiato il volto di questo Paese e dell'Europa, perché l'Italia esce dalla crisi economica più pesante dal dopoguerra ad oggi completamente cambiata, in quanto sono aumentate le disuguaglianze, le povertà, le marginalità, si sono avviati processi di vera e propria di desertificazione industriale, di deindustrializzazione; sono diminuiti drasticamente gli investimenti pubblici. Dal 2008 al 2018 gli investimenti pubblici sono calati del 46 per cento e solo nel 2018 il livello

che produca uno *shock,* di una politica economica e sociale che produca una svolta netta. Lo dico perché noi pensiamo (e lo abbiamo scritto anche nella nostra proposta di risoluzione) che non solo per noi non è un tabù superare i parametri imposti dall'Europa, o meglio quelli su cui anche il nostro Paese si è accordato all'epoca perché funzionassero, quindi il famoso livello del 2,4 per cento del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo; non solo non è un tabù arrivare a quel tipo di sforamento, ma pensiamo che quello debba essere il passo per cambiare davvero l'architettura delle regole e liberarsi di quella camicia di forza che la politica che la politica di *austerity* ha rappresentato in questa lunga stagione per i Paesi che invece avrebbero dovuto fare politiche di sviluppo. Tuttavia facciamo sommessamente notare che il Governo, che magari individua un tema importante, è molto lontano da questo obiettivo. tema è se volete cambiare il *fiscal compact* in sede europea e, se avete questa volontà, con chi avete intenzione di farlo. Lo dico per il suo tramite, signor Presidente, innanzitutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: se vi siete infilati in questa vicenda per cambiare quell'assetto con i Paesi di Visegrád, vi rivolgo i miei auguri perché quella è la direzione sbagliata e soprattutto è la peggiore. Per noi il tema non è

ossessionata dall'idea di capitalizzare quelle misure nei prossimi mesi in relazione all'appuntamento delle elezioni è una manovra nella quale emerge in modo palese una logica di tipo spartitorio. Intendo dire che quando ci si trova di fronte a una manovra nella quale ciascuna misura è perfettamente riconducibile a chi l'ha richiesta (in questo caso alle due forze che compongono la maggioranza), vuol dire che c'è una logica spartitoria e che manca un elemento principale, cioè lo sguardo strategico sul Paese, su dove si intende portare l'Italia dopo i lunghi dieci anni di crisi economica che l'hanno cambiata. Questo è ciò che noi pensiamo e lo diciamo perché all'interno delle misure previste ci sono aspetti positivi su cui non vogliamo aprire una discussione e un confronto. Penso ad esempio alla quota 100, anche se è immaginata in modo insufficiente e pasticciato, e al reddito di cittadinanza (di cui poi vedremo i contenuti), che assomiglia più a una misura di *welfare* compassionevole, anche con la supervisione di uno Stato etico che deve dire cosa consumare e cosa no. Insomma, sono misure su cui noi vogliamo confrontarci. Il tema è (lo dico ai colleghi della maggioranza): come fanno queste misure a stare insieme ad altre che hanno chiaramente un carattere regressivo? Voi vi accingete a preparare una misura che sta fuori dalla Costituzione, perché la *flat tax* (che è la misura Robin Hood al contrario, che toglie ai poveri per dare ai ricchi) sta fuori dalla Costituzione in quanto non rispetta la progressività fiscale. Come stanno insieme le misure sociali che voi avete individuato con la pace fiscale? Chiamatela per come la si dovrebbe chiamare, cioè un vero e proprio condono. condono. Questo è il punto di fondo. Per noi - e chiudo, signor Presidente - valgono alcune misure che dovrebbero essere prioritarie. Mettete un pezzo più consistente dell'extragettito sugli investimenti pubblici, innanzitutto nei settori strategici, nella manutenzione del territorio di un Paese che fa letteralmente acqua da tutte le parti (non è soltanto una metafora). Fate un'operazione diversa, altro che di pace fiscale e di *flat tax*;

la possibilità di immaginare una forma di tassazione sui grandi patrimoni, per fare politiche redistributive. Avete parlato di nazionalizzazione, all'indomani della tragedia di Genova, ma avete inserito in questo documento 10 miliardi di privatizzazioni. Volete spiegarci questa contraddizione? Se state sul piano delle rinazionalizzazioni in alcuni settori, noi vogliamo cercare un confronto. C'è poi poi un settore delicatissimo, forse il più delicato, quello del Sistema sanitario nazionale, la sanità pubblica. Avete scritto nero su bianco che questo Paese va

sotto quella soglia è un Paese che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, non può dirsi civile. Per questo - e chiudo davvero - noi pensiamo che si debba rimettere al centro questo tipo di priorità. Lasciate da parte l'ossessione per la prossima campagna elettorale e occupatevi di questo Paese, cosa che ci sembra non stiate facendo fino in fondo, perché state immaginando delle misure che non vanno nella direzione giusta e soprattutto che non fanno il bene di chi oggi ha pagato più di altri lo scotto della crisi economica.

dopo l'intensa serie di audizioni nei giorni scorsi è approdata in Aula la Nota aggiuntiva al DEF 2018, che contiene le linee programmatiche in campo economico che saranno alla base della prossima legge di bilancio. Durante le audizioni molti sono stati i rilievi e le preoccupazioni espresse dagli organismi auditi e da molti colleghi di minoranza (legittimamente, visto che è il loro ruolo), che considerano eccessivamente ottimistiche le previsioni degli effetti positivi di un'espansione della spesa capace di generare maggiori consumi, secondo stime - dicono - troppo discoste dalle linee tendenziali previste. interventi - lo dico per onestà intellettuale - sono stati importanti, di alto profilo e di stimolo a tenere sotto rigoroso controllo l'attuazione delle politiche avviate, permettendo, se necessari, precisi e tempestivi aggiustamenti correttivi. È vero che ogni Governo si trova davanti a scostamenti rispetto alle previsioni, come è stato detto durante le audizioni e come ha detto anche il ministro Tria: se saranno necessarie, si faranno. Aggiungo io: come altri Governi hanno fatto, mutate le condizioni. Alla luce comunque dei risultati degli ultimi anni, non si può negare che la crescita del PIL in Italia sia stata modesta (è stato ricordato in molti interventi che rimaniamo il fanalino di coda in Europa), così come la riduzione del debito non è stata molto significativa. Quindi rimaniamo convinti che occorra fare una manovra espansiva, come del resto stanno facendo altri Paesi in Europa, sforando l'obiettivo di *deficit* previsto. Ricordo le cifre: 2,4 per cento nel 2019, 2,1 nel 2020 e 1,8 nel 2021. Tanto per cominciare, per il 2019 il *deficit* al 2,4 per cento garantirà la disattivazione dell'aumento dell'IVA, che certamente potrebbe avere un effetto depressivo sui consumi, come temuto da tutti

Certamente, rispetto agli investimenti molti saranno gli stanziamenti, ma la grande sfida sarà trovare le

Questi giovani potranno costituire un patrimonio di risorse umane che cambierà le cose, grazie alla loro cultura moderna e aziendale e alla voglia di cambiare il mondo. Purtroppo, le generazioni

Dobbiamo riuscire a essere attrattivi verso questa generazione di intelligenze. Non solo, sono

macchina. Anche io sono un'amministratrice locale come il collega Zuliani. Pensate a quanto sono ingessati i Comuni, a quante opere sono rimaste bloccate e a quanto lavoro è stato fermato sarebbe potuto partire grazie alle opere piccole, medie e grandi delle migliaia di Comuni italiani. Fare oggi l'amministratore locale è una follia,

I Comuni sono ridotti all'osso e quotidianamente devono rispondere a quei poveri - e abbiamo capito che sono oltre 5 milioni - che bussano innanzitutto ai sindaci e agli assessori ai servizi sociali. Ci sono situazioni complicate,

i Comuni non sanno come fare per affrontare tutte queste emergenze. Allora dignità, fondi, velocizzazioni, ma se non parte il sistema anche a livello locale, non si va da nessuna parte.

una consulenza, dei servizi di assistenza con una professionalità altissima. Nelle Province, nei Comuni e in molti casi anche a livello di uffici statali non ci sono più professionalità così alte, e questo è un depauperamento. In questo senso le sfide sono davvero grandi, ma la linea tracciata c'è: è

per questo anno un'attenzione particolare ai piccoli, perché un alleggerimento possa permettere ai piccoli di ripartire e di assumere;

e siamo sicuri che la loro vita è il lavoro, perché il lavoro è dignità; c'è una cultura del lavoro. Quindi questi soldi non saranno sprecati, ma creeranno

con attenzione, non da irresponsabili perché abbiamo dei ruoli che non ci consentono di essere irresponsabili; con prudenza, ma anche con coraggio e lo faremo convintamente guidati dai nostri Ministri e dalla nostra squadra di Governo.

negli interventi precedenti il DEF è già stato scavato, difeso e abbondantemente criticato. Mi limiterò a costruire una cornice dei rischi nei quali l'Italia potrebbe sprofondare nell'arco delle prossime settimane, in ragione di tre fattori che questa mattina, da parte della maggioranza e di chi sostiene il Governo, non sono stati assolutamente contestati. Vedo la debolezza di questo Documento soprattutto in tre fattori. La conferma di scarsi investimenti: ieri ne abbiamo discusso in Commissione infrastrutture e trasporti. La cifra complessiva non è assolutamente in grado non dico di favorire una forma di qualsiasi crescita di questo straordinario Paese, ma non ma non è nemmeno in grado di portare a conclusione impegni presi nel campo infrastrutturale dai Governi che hanno preceduto l'attuale Il secondo fattore da sottolineare è che vi è una netta prevalenza di interventi di natura redistributiva: e lì ci fermiamo. Il terzo è che, scavando nelle tabelle del Documento di economia e finanza, è assolutamente impossibile rintracciare una qualsiasi sottolineatura che riguardi la scuola e la cultura. E senza evidenze di investimento di fondi in scuola e cultura è difficile costruire un futuro

costruiscano uno scenario deleterio grazie a questa manovra, facendo sprofondare l'Italia a un livello più basso della tripla B attuale, è un rischio che non possiamo permetterci e consentire. Non fosse altro perché esistono perché esistono molti istituti di credito e di investimento europei, a cominciare da quelli svedesi e da quelli tedeschi, che hanno nei loro statuti l'obbligo a non investire in Paesi considerati, se scendono di livello, Paesi spazzatura. L'opinione che ci si sta formando per i titoli di Stato italiano è che, se non si ricorre a una sorta di manovra da oro alla Patria della fine degli anni Venti, l'Italia non abbia più un attaccapanni reale dove appendere una parte rilevante del proprio debito. C'è una considerazione da fare, perché mai immagino che chi si trova a governare un'Italia così straordinaria sia

per costruire uno scenario che è avulso dalle nostre radici, lontano dalla nostra identità e che si appresta a costruire una cornice europea decisamente diversa da quella che abbiamo conosciuto. Lo scontro oggi, signor Presidente, non è più tra società aperta e società solidale. Lo scontro in Europa e nel mondo oggi è fra società aperte e società solidali, da una parte,

e vivo questa storia con preoccupazione. Noi oggi viviamo la prova generale di questa storia. Questo è il primo vero provvedimento del Governo, ben più ancora delle misure sui migranti, che traccia questo fossato. Non è una linea di confine, ma una frontiera difficilmente valicabile per chi crede che società aperta e società solidale possano ancora oggi esistere.

oggi siamo qui a discutere della Nota di aggiornamento al DEF presentata dal Governo, che fissa le linee per la prossima legge di stabilità. Una Nota, a nostro parere, superficiale e dalla quale (sono molti i casi) non si intuiscono le modalità degli interventi annunciati. Vedete, a noi non spaventa una manovra in *deficit*. Ogni buon padre di famiglia nella sua vita ha deciso di indebitarsi per raggiungere obiettivi importanti: l'acquisto di una casa, le cure odontoiatriche per i propri figli, l'avvio di una nuova attività. Debiti sempre finalizzati ad un miglioramento della qualità di vita. Miglioramenti che, invece, facciamo fatica a trovare nella Nota. Questa Nota non ci dà grandi speranze, ma una unica certezza. Dopo il varo della manovra gli italiani acquisiranno un maggior debito *pro capite*. Per entrare nel concreto, avremmo voluto un'introduzione più decisa della *flat tax*; avremmo voluto più sgravi alle imprese che assumono i giovani, che appaiono essere dimenticati nel Documento oggi in discussione. Avremmo voluto che, prima di impegnare 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, si fosse pensato al mondo della produzione, a chi i posti li crea per davvero e non li racconta. Un reddito di cittadinanza che sapete benissimo non partirà subito, perché si basa sulla riorganizzazione dei centri dell'impiego, che oggi sono un buco nero, non funzionano: i dati raccolti ci dicono che solo il 3,2 per cento degli iscritti ai centri per l'impiego ha trovato una risposta. Voglio ricordare anche che dal 2003, con la legge Biagi, anche i privati e altre istituzioni come ad esempio le università possono svolgere le stesse mansioni dei centri per l'impiego, ed allora la domanda nasce spontanea: non era forse il caso di verificare anche i dati di queste organizzazioni per capire la situazione dell'offerta lavorativa, prima di pensare ad un forte investimento sui centri per l'impiego? quindi con forza che, prima di assumere migliaia di persone per i centri per l'impiego, si doveva procedere nell'aiutare le imprese a creare occupazione, per generare un incremento dell'offerta lavorativa. Meno tasse, sgravi per le aziende, incentivi alle nuove assunzioni: questo doveva essere il filo conduttore della manovra. Per restare sempre nel tema del reddito di cittadinanza, ci sono interventi già sperimentati ed ancora attuali come il REI, che di fatto si sta rivelando un mero intervento assistenzialista per mancanza di offerta dal mondo del lavoro. E voi che fate? Ne aggiungete un altro. So che non prenderete in considerazione le nostre osservazioni, perché questo è un provvedimento che in termini elettorali ha un suo valore, eccome se ce l'ha. Ma andiamo avanti. L'occupazione giovanile - tema delicato ed emergenziale nel nostro Paese - trova cittadinanza nella Nota esclusivamente nell'utilizzo dello sblocco del *turnover* nelle pubbliche amministrazioni. Tutto qui? Ci sembra veramente poco. Arriviamo al tema pensioni, argomento che ci sta a cuore. La quota 100 era nel nostro programma, ma vorremmo meglio capire cosa intendete quando parlate di pensione di cittadinanza. Se l'intenzione è di portare a 780 euro la pensione di chi oggi percepisce la pensione sociale che ammonta a poco più di 400 euro, va bene, ma contestualmente devono essere aumentate a 1.000 euro le pensioni minime. Per noi la differenziazione è sostanziale, perché chi percepisce la pensione sociale non ha mai versato un contributo, a differenza dei percettori delle minime, che li hanno sempre versati. Sulla disabilità e gli anziani, accogliamo con favore l'aumento del fondo per la non autosufficienza, che negli anni ha subito molti tagli e che di fatto sta rendendo difficilissima la gestione assistenziale degli anziani. Altrettanto dicasi per l'incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che speriamo sia consistente per l'avvio di progetti di vita indipendente e di tutoraggio all'interno delle aziende che assumono persone con disabilità. Dopo le note positive appena descritte, però, ci saremmo aspettati di trovare almeno un accenno ai lavoratori precoci, che saranno penalizzati da quota 100. Nemmeno una parola sul dopo di noi, sui *caregiver* all'interno della Nota. Nota che dice di voler incentivare gli interventi sulla domiciliarità e poi ignora questi argomenti perde di credibilità. In conclusione, il Documento presentato appare evidente che sia frutto del contratto di Governo

ed è così che in queste ore mi sono ritrovato ancora una volta con «Lehman Trilogy», scritto da Stefano Massini. Ve lo consiglio, è un libro interessante, perché guarda caso arriva a dieci anni dal fallimento di un paradigma, quel paradigma la cui eco si ripercuote ancora in queste ore in cui si parla di *spread*, in cui si torna a rimasticare gli stessi lemmi che avevamo un po' dimenticato dieci anni fa. perché il mondo crollò dieci anni fa, il fallimento della Lehman è esattamente del settembre di dieci anni fa. Quella dovrebbe essere la lezione per capire che coloro che avevano previsto, visto, ma anche un po' creato quel bubbone sapevano già tutto, ma facevano finta di non saperlo. E chi erano gli attori protagonisti di quel bubbone? Erano gli stessi che oggi ci dicono che è prevista la tragedia.

Lehman Brothers insieme ad altre banche d'affari. Allora fallì Lehman Brothers, ma il giorno precedente Bank of America salvò Merrill Lynch e poche ore dopo furono costretti a salvare AIG, il colosso assicurativo. Eppure, tutte le agenzie di *rating* e tutto l'esercito di professoroni ed economisti continuavano a dire «Va tutto bene, Madama la marchesa». Perché preoccuparsi? Ebbene, gli stessi soggetti oggi ci dicono che forse domani sarà la tragedia, forse domani. Commentiamolo oggi. Commentiamo le macerie che questo sistema ha visto crollarsi addosso e in qualche modo subire. La crisi che stiamo vivendo è una crisi non economica,

a chi ieri ha fallito, a chi ieri diceva che la finanza in quelle banche d'affari era troppo grande per fallire, era un sistema troppo perfetto per fallire e invece gli è caduto addosso. Ed è quel crollo ad aver provocato la crisi cui oggi cui oggi dobbiamo fare fronte. Ecco perché fino adesso, dieci anni dopo, abbiamo assistito sempre alle stesse dinamiche per cui le manovre finanziarie del passato avevano scommesso sull'austerità.

a riflettere sulle dinamiche finanziarie che ancora oggi ci sono proposte come un modello di riferimento. Mi rivolgo anche ai colleghi giornalisti che

Allora varrà la pena di domandarsi se una qualche protezione non dovrà venire da Bankitalia, sempre che essa sia ancora alleata del sistema Italia. Ultima considerazione: la manovra deve la manovra deve guardare all'economia reale. Arrivo da un confronto con alcuni lavoratori, ce ne sono tanti e ogni giorno facciamo i conti con crisi aziendali. Quando i lavoratori arrivano sul tetto, a lamentarsi e protestare perché qualcuno viene licenziato perché non è fedele

PD)*. Io credo che il senatore Paragone farà carriera nel MoVimento 5 Stelle, perché la possibilità di fare carriera nel MoVimento 5 Stelle è direttamente proporzionale al numero di corbellerie che si sparano.

Non pensavo, però, potessero andare oltre, né Paragone, né Di Maio La Qualunque. Pensavo che fosse impossibile

Noi abbiamo superato però il limite anche rispetto a questo. Poco fa il ministro Lezzi ci ha deliziato con i condizionatori e il PIL e io pensavo che anche questo fosse insuperabile. Invece ieri in Commissione salute ho avuto la possibilità di ascoltare il sottosegretario alla salute Bertolazzi, cui poi è andato in soccorso il senatore Endrizzi,

quale, lo scienziato (che diventerà ministro sempre per quella teoria che più ne spari, più vai avanti) ci ha spiegato che con il reddito di cittadinanza, di fatto, noi contribuiamo a finanziare la salute, perché i cittadini pagheranno con quel reddito anche le spese mediche.

Questa è la modalità con la quale viene costruita una manovra che riguarda il futuro dei cittadini. Non ci sono risorse effettive. Ci sono sono risorse che vengono utilizzate soltanto prendendo i soldi dal futuro delle nuove generazioni, e quindi l'indebitamento, con l'idea di trasformare il Mezzogiorno in una casa di riposo, in modo che la Lega

crediamo che stiate portando il Paese al fallimento e le nuove generazioni nel baratro.

abbiamo avuto occasione di ascoltare tutti gli interventi, molti dei quali forse non ne tengono conto - che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza è sostanzialmente una cornice programmatica. Prima di criticare le misure bisognerebbe forse aspettare che vengano declinate nella manovra.

parte di altri attori a livello europeo, e non solo. Rispetto al passato, possiamo dire che, finalmente, abbiamo un Governo che mette nel Documento di economia e finanza un rapporto *deficit*/PIL che,

che 1,8; poi arriva l'ISTAT a fine anno e dice che siamo al 2,4. Meglio, quindi, essere chiari fin dall'inizio e rispettare quello che si scrive nei documenti, sembrano piuttosto artifizi per far passare la manovra e far capire che è tutto a posto, salvo poi, quando si va a vedere a consuntivo i conti, rendersi conto che le cose sono un po' diverse rispetto a quelle programmate. Abbiamo messo in evidenza con grande chiarezza due elementi chiave che accompagnano la Nota di aggiornamento: responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, che sono, naturalmente, dettati dal seguente fatto. Se è pur vero che è sbagliato dire che ci avete consegnato un Paese al disastro - non è vero, non sarebbe corretto e non sarebbe assolutamente giusto - è altrettanto vero che non si può neanche dire che ci avete consegnato un Paese che stava andando a gonfie vele e si stava riprendendo. *(Applausi dai Gruppi è l'ultimo dei Paesi europei, significa che non siamo allo sfascio, ma non siamo neanche i primi della classe; anzi, a dire il vero, siamo proprio gli ultimi. Proprio per questa ragione occorre

alla fine i soldi ci sono, ma in Italia si fa fatica a spenderli. Certo, se facciamo come in passato e concentriamo gli investimenti su nuove opere da realizzare, avete ragione voi: di sicuro fra cinque anni saremo ancora qui punto e a capo - ahimè, lo dico - e dall'altra parte il Prodotto interno lordo non si muove neanche di una virgola. una novità in questa Nota di aggiornamento, ossia che, a differenza del passato, gli investimenti saranno concentrati soprattutto sulla sistemazione dell'esistente, che da un punto di vista culturale

i ponti, e poi il Paese si deteriora. Facendo investimenti di questo tipo e ristrutturando l'esistente, non penso che occorrano particolari permessi, tutta una burocrazia; ci vuole poco. E, quindi, questo vuol dire mettere subito in campo energia per così dire positiva: le

che - vivaddio! - hanno governato e amministrato bene, visto che hanno messo un po' di fieno in cascina, come dalle nostre parti si usa a fare quando bisogna amministrare e pensare alla propria famiglia.

che le stime della nostra Nota di aggiornamento siano davvero prudenziali, perché crediamo che il Paese crescerà di più rispetto a quanto è stato scritto, e non di meno, come i tecnici e i burocrati vogliono farci credere.

persona che andrà in pensione in modo anticipato, sia possibile assumere uno o due giovani, perché alla fine comunque l'azienda manderebbe fuori dal mercato del lavoro un lavoratore che costa parecchio e ne potrebbe inglobare uno che costa molto meno, il fatto di creare posti di lavoro non è una misura o uno stimolo alla crescita?

«Caspita, questi qui del Governo giallo-verde, legastellato o populista-sovranista - chiamatelo un po' come volete - chissà mai che riescano davvero a cambiare la legge Fornero e poi magari a dimostrare che il sistema sta in piedi lo stesso?». Cosa vorrebbe dire questo? Vuol dire sconfessare tutto quello che negli ultimi sette anni ci avete raccontato. Questa è la paura che avete voi che avete fatto quella legge e l'avete votata, e noi sappiamo bene chi ha votato quella legge.

lo dico a beneficio di tutti - se la manovra la devono fare i mercati, allora domani mattina andiamo tutti a casa, perché vuol dire che qua non serviamo a niente non serviamo a niente e siamo stati eletti per niente: questa è la verità e dobbiamo capirlo bene.

gli interessi dei cittadini italiani? Io non ci credo assolutamente e, anzi, penso sia giusto rispettare le regole e stare nella legislazione. Ci mancherebbe altro, perché la sovranità appartiene al popolo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione,

l'Italia sarebbe nella media e, invece, la Francia, tanto osannata, sarebbe tra gli ultimi posti. *(Applausi

preoccupati ma anche speranzosi per quanto succede in quest'Aula dove, senza enfasi ma con orgoglio, non ho difficoltà a dire che, per la prima volta, dopo troppi anni, si mette in campo una manovra economica

fare con grande forza ciò che tutti i manuali di politica economica insegnano e tutto ciò che è tra le aspirazioni principali dei politici come noi, che, in quest'Aula, oggi affrontiamo argomenti tanto delicati: avere a disposizione risorse adeguate non solo per soccorrere le emergenze, ma anche per spingere in un clima di fiducia generale l'economia verso la crescita, facendo magari schizzare in alto quegli indici economici che banche e grandi investitori guardano con attenzione quando devono investire in fiducia e in risorse in un Paese piuttosto che in un altro. Ho l'orgoglio questa mattina di plaudire una manovra economica che, per la prima volta, dopo tantissimi anni, mette in campo delle idee e delle risorse per fronteggiare i problemi principali del Paese. In campagna elettorale di avere grandi ambizioni di Governo per rimettere a posto l'economia del Paese e per ridare fiducia alle famiglie. Gli italiani con grande fiducia ci hanno votato, come nessuno magari sperava e si augurava, e noi oggi siamo qui per fare quello che abbiamo promesso ai cittadini, con la fiducia e la sicurezza, però, di chi ha l'occhio attento ai conti pubblici, alle compatibilità e - perché no - anche al rispetto dei trattati internazionali. Tuttavia - come capita a chi sinceramente si vuole cimentare con i problemi più importanti di un Paese in grande difficoltà, e l'Italia ha conosciuto tante e troppe fasi di questo tipo - quando arrivano al Governo forze autenticamente riformiste,

gli italiani si aspettano tanto dalla classe politica - e da noi in particolare per gli impegni assunti ma hanno ormai la coscienza, come tutti noi dobbiamo avere anche quando critichiamo questa manovra, che siamo con le casse pressoché vuote. Ci è stato consegnato un Paese in cui ci sono milioni e milioni di cittadini sotto la soglia della povertà e tutto questo in uno dei Paesi occidentali considerati più sviluppati. Parliamo di milioni sotto la soglia della povertà; famiglie che non riescono più a far studiare i propri figli; giovani che non riescono più a studiare o che, dopo aver studiato, devono emigrare perché non ci sono risorse. Di chi è la colpa di tutto questo? tutto questo? È una responsabilità storica e dovrebbe ricordarsene chi oggi con troppa facilità, dopo aver governato il Paese, si permette di criticare dimenticando ciò che ha fatto, non un secolo fa, ma solamente negli anni scorsi per ridurci in tale situazione. Per questo dico che la manovra economica deve essere rivendicata con orgoglio dalla maggioranza di Governo e deve arrivare ai cittadini anche con il racconto giusto.

per i commentatori, per i giornalisti, per tutti i giornali e per tutte le televisioni. Nella mia vita ho fatto il giornalista e so quanto è prezioso il bene dell'indipendenza, soprattutto perché siamo in un Paese

ricordando però che sarebbe importante guardare sempre ai dati e alle cifre senza posizioni preconcette. Noi non vogliamo non vogliamo giornalisti amici. Noi vogliamo solamente buon giornalismo in Italia e un racconto obiettivo di quello che capita in questo Paese. È fondamentale allora che ci sia un racconto giusto e obiettivo di quello che stiamo facendo perché, dinanzi alla situazione disastrosa che stiamo fronteggiando in questo momento, che è l'eredità che un'intera generazione di politici e soprattutto gli ultimi Governi ci hanno consegnato, mettiamo in campo una manovra che ha l'ambizione di porre mano e fronteggiare le due emergenze del Paese. C'è innanzitutto l'emergenza sociale, e non voglio ripetermi sulla povertà e sulla situazione disastrosa di milioni di cittadini che non hanno letteralmente più i mezzi per vivere. Lo facciamo mettendo in campo quel reddito di cittadinanza che non è un atto d'avventura, ma è solamente la misura minima che un Parlamento solidale deve in questo momento ai cittadini che ci ascoltano e che non sanno come arrivare a fine serata Mettiamo in campo una misura cosiddetta di pensione di cittadinanza che porta a un reddito minimo, quello della soglia di povertà, le pensioni cosiddette minime. Tale intervento non scardinerà certo i conti dello Stato - come voi tutti sapete bene - ma è un atto elementare di solidarietà che una classe politica in grande debito con

segua attentamente il mio intervento - sarà con me nel dire che le pensioni di cittadinanza a 780 euro non scardineranno certamente i conti dello Stato.

di mettere in campo le risorse necessarie per spingere i settori trainanti dell'economia. Ci sono

sono gli investimenti pubblici a far ripartire le economie agonizzanti. Ci avete lasciato solamente la possibilità di investire 15 miliardi, ma noi li rivendichiamo come un tesoro perché, al di là delle cifre, sono un segnale preciso di un'inversione di un'inversione di politiche economiche che, per la prima volta in Italia, cercano di dare una prospettiva di crescita all'economia del Paese.

per andare a reperire anche le decine di milioni appostati in settori parassitari per spese che non servono a questo Paese per immetterli nel ciclo virtuoso di investimenti. signor Presidente, richiamando anche lo sforzo che stiamo facendo per sbloccare un autentico tesoro costituito da quei 150 miliardi annidati nei meandri della pubblica amministrazione, frutto del patto di stabilità, di tutte le pastoie le pastoie imposte alle amministrazioni locali negli ultimi anni, per tirar fuori anche da lì le risorse necessarie alle altre emergenze che ci avete maledettamente lasciato. Con quei soldi spero e sono sicuro che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali ci aiuteranno a mettere mano a tutte le altre emergenze che ci avete lasciato. alle emergenze sismiche, con il 90 per cento delle scuole di questo Paese vergognosamente prive dei necessari requisiti di sicurezza, che - tradotto tutto in parole povere - vuol dire che i precedenti Governi in questo momento mettono le famiglie nella condizione disperata di mandare nelle scuole nelle scuole i propri figli con il rischio che i tetti, in caso di sisma (ma non solo), gli piovano in testa. Questi sono i due obiettivi della manovra. Sono obiettivi chiari, chiari, che contengono anche il messaggio che questa maggioranza e questo Governo, con grande tranquillità, lanciano ai cittadini e ai cosiddetti mercati e alle istituzioni europee, perché sono un segno di grande fiducia per il nostro Paese: fronteggiamo le emergenze della povertà

di estrema povertà, che riceveranno il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza. Per questo dico, e vedete con quanta tranquillità lo faccio... PRESIDENTE. Non credo, per le cose dette, che ci sia da allarmarsi più di tanto, né può far testo la preoccupazione dell'Ufficio parlamentare parlamentare di bilancio. Noi siamo tranquilli e i conti dello Stato sono al sicuro. Da qui oggi parte un messaggio ambizioso per il futuro del Paese, ma anche di estrema tranquillità per chi ci ascolta e deve allocare le proprie risorse, che sono i risparmi personali o i depositi dei risparmiatori. *(Applausi

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto mi sia consentito di osservare una contraddizione. C'è stato un grande dibattito in quest'Aula, qualche tempo fa, a proposito del decreto dignità. dignità. In quel decreto-legge si mettevano all'indice il gioco e le scommesse; ebbene, ora si punta tutto sulla scommessa che il prodotto interno lordo italiano possa crescere oltre le più ottimistiche previsioni. Nessuno degli istituti nazionali e internazionali ha stime di crescita come quelle inserite in questa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Oltretutto, vengono rassegnate previsioni di crescita più ottimistiche in presenza di un quadro internazionale in deciso peggioramento, che aveva indotto a rivedere al ribasso, da parte di questo Governo, le previsioni a legislazione vigente; il tendenziale è stato corretto in negativo e non in positivo. La progressione del prodotto interno lordo programmatico, qualora si avverasse, potrebbe portare a circa 2.000 miliardi di prodotto interno lordo italiano nel 2022. Viene infatti aumentato a 1.816 miliardi nel 2019, l'1,5 per cento e 6,6 miliardi in più rispetto al valore tendenziale (un primo anno ritenuto dalla maggioranza prudente);

nel 2021, portando quindi il prodotto interno lordo a 1.946 miliardi, quindi vicinissimo ai 2.000 miliardi. Sulla base di queste stime, migliora anche il rapporto tra debito e PIL.

Il rientro del *deficit* verso l'obiettivo europeo è ovviamente rallentato, basandosi almeno la metà della manovra sul maggior indebitamento. Sulla crescita il Governo punta proprio tutto, perché solo un aumento del denominatore può ricondurre a parametri accettabili il rapporto tra debito e PIL.

Quindi, siamo in una condizione lontanissima dai valori di crescita dei Paesi che sono i primi in Europa e a cui le nostre imprese non hanno peraltro nulla da invidiare e con cui sono in piena competizione. Recuperare questo *gap* nella crescita sarebbe un fatto auspicabile da tutti, compresi noi, che siamo un'opposizione responsabile. Questo è l'augurio che noi facciamo all'Italia, prima che al Governo. Quello che ci chiediamo è se le misure annunciate siano adeguate a innescare un autentico *shock* nella crescita, che nessuno dei moltiplicatori utilizzabili può al momento far presagire. Manca infatti una decisa riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi.

consentitemi di dire assistenziali, ma non in senso denigratorio, come quelle previste per il reddito cittadinanza e le pensioni, attraverso l'aumento della minime e l'introduzione di quota 100.

La letteratura economica e la prassi ci insegnano che - ahimè - nella storia hanno sempre avuto moltiplicatori abbastanza bassi,

La crescita potrebbe essere innescata da disposizioni in deroga alla miriade di vincoli che frenano l'utilizzo dei fondi europei (vorrei ricordare i più di 50 miliardi della programmazione 2014-2020, riguardanti gli investimenti, che sono fermi in questo Paese), oppure in deroga alla pletora di norme e cavilli che vincolano gli investimenti sulle infrastrutture nonostante gli stanziamenti siano già previsti. Stiamo parlando di 100 miliardi di euro, quindi una cifra ben superiore ai 15 miliardi nel triennio citati in alcuni interventi. È apprezzabile l'aggiunta di 15 miliardi nel triennio, ma ritengo che il Governo debba sbloccare e investire i 100 miliardi già stanziati.

Siamo sicuri che un Governo in cui l'azionista di maggioranza si è sinora espresso in sintonia con No

Siamo sicuri che coloro che hanno sinora agitato le manette possano ammettere procedure che velocizzino i passaggi per realizzare le opere pubbliche? Sono domande che vi rassegno, sperando in una risposta positiva, per il bene del nostro Paese, perché le conversioni sono sempre le benvenute. Certamente, se l'altro azionista della Lega in questo Governo fosse Forza Italia, non avremmo dubbi che gli investimenti, specie in infrastrutture, sarebbero partiti e sarebbero stati sostenuti tutti.

Ora, il cosiddetto decreto Genova pare non crei le stesse condizioni. «In deroga a», e segue un elenco di norme, ma in buona sostanza tutto rimane fermo, perché oltretutto negli ultimi anni è stato anche appesantito il codice degli appalti.

che non ci sono. Noi crediamo che una manovra che punta sulla crescita sarebbe credibile se fosse proposta da un Governo in cui ci fosse un partito molto meno statalista e un po' meno pseudo-ambientalista. È un Movimento che dice tante cose che piacciono alla gente, ma le cui contraddizioni ideologiche sono talmente tante da non riuscire a risolvere nessuno dei problemi anche nelle città che governa. Guardiamo il caso di Roma Capitale: dopo due anni è emblematico, funziona solo il servizio di transennamento. Guardate Torino sulla via della decrescita felice, fabbrica di disoccupati. Noi, ovviamente, speriamo vivamente di sbagliarci e che ci sia la crescita auspicata. Nella nostra risoluzione sono inseriti molti punti, d'auspicio, d'augurio, e speriamo accoglibili. Non dimenticatevi mai una cosa: che noi tifiamo, sempre e comunque per l'Italia. Peraltro ci chiamiamo Forza Italia.

il Governo con la Nota di aggiornamento al DEF compie il primo passo per un'importante opera di rinnovamento del nostro Paese; lo fa iniziando dalla tutela dei cittadini più deboli e maggiormente colpiti dalla crisi e dallo *stop* alle politiche di austerità

rafforzamento del *ventures capital* del piano Impresa 4.0, promozione dell'innovazione tecnologica e tutela delle piccole e medie imprese. Al contempo, vengono realizzati due importanti interventi di sostegno a lavoratori e famiglie: il reddito di cittadinanza e quota 100. Si tratta di due misure di civiltà giuridica che aiutano i cittadini più deboli. Il reddito di cittadinanza aiuta coloro che si trovano, a causa della crisi, in condizione di marginalità sociale e, al contempo, permette di sostenere e rilanciare l'economia attraverso i consumi. Quota 100 è una misura che consente il ricambio generazionale liberando posti di lavoro, garantendo quindi attraverso un adeguato *turnover* l'ingresso nel mondo del lavoro di manodopera giovane, qualificata e con una elevata propensione all'innovazione. Abbiamo ovviato alla rigidità che la legge Fornero aveva introdotto, superando un impianto previdenziale rigido e penalizzante per i lavoratori. Dopo anni di strenue lotte, finalmente l'attuazione del reddito di cittadinanza è realtà grazie alla tenacia, alla coerenza e all'impegno del nostro Movimento. Il reddito di cittadinanza non consiste - per chiarirlo ai colleghi - unitamente in un'erogazione monetaria di 780 euro al singolo, ma è una misura proattiva di reinserimento nel mondo del lavoro che coinvolge l'intero nucleo familiare. Non si tratta di elargire un sussidio incondizionato, ma di concedere un doveroso aiuto in cambio di un impegno reale e attivo nel reinserimento sociale e nella ricerca del lavoro. Formazione, lavoro per la comunità,

è strettamente collegata ad esso la riforma dei centri per l'impiego, che verranno notevolmente potenziati e riorganizzati, sia in termini di risorse umane sia in termini di infrastruttura tecnologica. I centri per l'impiego devono diventare il canale principale di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Perché ciò possa realizzarsi è necessario intrecciare e interconnettere tutte le banche tutte le banche dati esistenti. I centri per l'impiego sono il primo passo verso la digitalizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni, che devono operare in maniera sinergica, agevolando il cittadino e semplificando pratiche e procedure burocratiche. Proprio per questo tecnologie innovative, come la *blockchain*, potranno giocare un ruolo determinante nel rinnovamento e nella digitalizzazione del nostro Paese. Il programma illustrato nella Nota di aggiornamento al DEF pone un'attenzione particolare anche a chi, pur percependo una pensione, si trova comunque al di sotto della soglia di povertà relativa. Si tratta soprattutto di donne e lavoratori precari che hanno avuto una carriera discontinua. La misura che viene introdotta dal Governo consiste in un'integrazione della pensione percepita, fino al raggiungimento di 780 euro per il singolo. Si tratta di un aiuto concreto che permetterà di ridare dignità a migliaia di cittadini italiani. Per concludere vorrei fare, signor Presidente, delle riflessioni. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi in quest'Aula e mi è sembrato molto singolare ascoltare interventi che andavano a richiamare la Costituzione italiana, ma parlando solo ed esclusivamente di un articolo, ovvero dell'articolo 81. Io ricordo a tutti noi e a quest'Aula che ci sono dei princìpi fondamentali che sono inseriti nella Costituzione italiana: a partire dall'articolo 2, dall'articolo 3 e dall'articolo 36, che sono oggetto delle nostre riforme e di quanto il Governo, questo Governo, ha inserito nel DEF. Questi sono i nostri intendimenti. Vorrei allora fare una riflessione con i colleghi e pensare che, forse, è il caso di mettere per la prima volta al centro della politica di Governo e di tutti i parlamentari presenti, in quanto rappresentanti dei cittadini italiani,

e a chi ha governato precedentemente a noi che il Mezzogiorno è stato abbastanza dimenticato. *(Applausi dal quando si parla di sgravi contributivi e di aiuti al Mezzogiorno, che il *jobs act* a nostro parere ha poco influito sull'occupazione vera in Italia, se non sui dati sulla disoccupazione; se siamo tra i Paesi con i salari più bassi in Europa e se aumenta ancora la soglia di povertà e il numero di famiglie povere, è chiaro che il dato sull'occupazione va guardato nella sua completezza. Voglio poi ricordare a tutti in quest'Aula, e chi c'era lo sa, che il *jobs act* è stato finanziato sopprimendo proprio uno sgravio contributivo che era destinato agli imprenditori del Mezzogiorno, che era una misura strutturale, non soggetta

non parziale, ma completa. Noi abbiamo già messo fine alla precarietà con il decreto dignità e abbiamo iniziato ad aiutare le aziende.

è un investimento che Paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo hanno già messo in atto. Questi sono gli investimenti per il Paese. Ci è stato detto che non sanno cosa accomuna la Lega e il MoVimento 5 Stelle. Io ho scritto la risposta: ci accomunano ci accomunano la grande vicinanza con il territorio, il legame con i cittadini e con le loro esigenze, il rispetto degli impegni presi e la volontà di cambiare

sulla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, la proposta di risoluzione n. 100, presentata dai senatori Patuanelli e Romeo.

Signor Presidente, membri del Governo, senatrici e senatori, limiterò ad una breve replica, non potendo entrare nel merito di tutti gli interventi svolti dalle colleghe e dai colleghi, che ho ascoltato con molta attenzione, rilevando punti negativi ma anche punti positivi. Ovviamente, replicherò a quelli negativi. I concetti che sono stati espressi vertono quasi tutti sulla preoccupazione che questa NADEF possa non raggiungere l'effetto sperato, ma allo stesso tempo ho potuto leggere tra gli interventi un senso di necessità che si debba cambiare passo e che molti degli aspetti toccati da questa NADEF, ossia il supporto a chi è uscito dal circuito del lavoro o non vi è entrato (con il reddito di cittadinanza), il supporto al ricambio generazionale con il superamento della legge Fornero, le intenzioni e gli importi decisi dal Governo in merito agli investimenti siano tutti obiettivi condivisi dal quasi intero arco parlamentare, in forme e tempi sicuramente diversi ma condivisi. Altre preoccupazioni emerse dal dibattito sia in quest'Aula che in Commissione bilancio vertono sui tempi di ottenimento dei benefici di questa manovra. Si è detto che dodici collegati sono troppi e non ce la si farà a metterli in atto in pochissimi mesi, ma voglio sottolineare che tutte queste sono azioni che ci rimettono in linea con il resto dell'Europa e quindi vanno portate avanti e non possiamo che agire su questo binario, visto che le manovre effettuate in questi ultimi anni non ci hanno fatto crescere che di miseri punti percentuali prossimi all'unità. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che gli investimenti possano non dispiegarsi con i tempi giusti a causa della burocrazia elevata, ma nella NADEF sono previste azioni proprio volte a semplificare e a ridurre la burocrazia e a creare cabine di regia per rendere più veloci i processi (proprio ieri si è tenuto il primo incontro a Palazzo Chigi). In merito al Sud, al fatto che non viene praticamente citato nella manovra, io sono di Bari e a questo punto non posso sottrarmi dal replicare (mi dispiace sia assente la senatrice Bellanova). Siamo lieti che l'attenzione al Mezzogiorno e l'invito alla coesione territoriale vengano da una rappresentante eletta in Emilia-Romagna e ricordo che abbiamo un Ministro per il Sud che viene proprio dalla terra di Lecce (che poi è anche la terra della senatrice Bellanova), e non c'è bisogno di indicare misure specifiche in manovra, perché il Ministro sta attivamente lavorando con tutti i presidenti di Regione proprio per far sì che i fondi di coesione spesi in questi anni in maniera poco efficiente (ricordiamoci i progetti sponda), ma soprattutto quelli non spesi possano essere utilizzati in maniera efficace ed efficiente, in modo da dare un effettivo rilancio al Sud. Si è detto che non si potrà riuscire a vendere gli immobili dello Stato per l'ammontare inserito nella misura perché in passato non vi si è mai riusciti. Ma se da un lato è vero che la storia del passato indica la via, dobbiamo pensare al futuro in maniera diversa e non è detto che, siccome in passato non si sia riusciti, questo debba essere vero anche per il futuro. Sia ben chiaro che questo Governo non intende depauperare il patrimonio: intende vendere gli immobili che non servono più allo Stato; non intende quindi fare favori a chicchessia. Se continuiamo a guardare al passato, l'Italia non si risolleverà e noi, ma noi tutti, non solo questa maggioranza, saremo condannati a essere soltanto testimoni del declino senza poter fare alcunché, invece siamo qui proprio per dar vita al cambiamento. Si è detto che la manovra indebolisce la credibilità del Paese perché il quadro previsionale non è stato condiviso da Istat, Corte dei conti, Banca d'Italia e non è stato validato dall'UPB. Al contrario però dobbiamo pensare che proprio perché questa manovra è completamente diversa dalle precedenti manovre (che ci hanno portato - vorrei ricordarlo - esattamente qui dove siamo, con il risultato del 4 marzo), i mercati, soprattutto quelli esteri, la approveranno perché si renderanno conto che l'Italia ha deciso di cambiare passo, di fare quel cambiamento che è anche il marchio di fabbrica del Governo. Il Presidente del Consiglio e i Ministri hanno cominciato ad incontrare istituzioni e operatori dei mercati esteri proprio per illustrare la manovra, perché i soli numeri talvolta non riescono a rendere bene la portata delle modifiche. Qualcuno ha detto che questo Governo non ha un disegno. Credo invece che nella NADEF sia ben delineato il disegno in grado di cambiare le sorti dell'Italia. Questa manovra è espansiva e non di *austerity* come le precedenti. Pertanto è più che comprensibile che i colleghi, molti dei quali presenti in quest'Aula da più legislature, abituati ad altri tipi di manovre, si possano sentire a disagio nell'accettare una così forte quantità di cambiamenti e sentano la pressione della possibilità che tali cambiamenti, che pur condividono, possano non avverarsi. Lo stesso disagio è provato dai vari enti che non si sono espressi positivamente sulla manovra perché abituati ad analizzare manovre recessive e perché i modelli utilizzati tendono a dare eccessivamente la precedenza alla prudenza, con il rischio anche di abbattere le parti positive presenti nelle manovre. Vorrei ricordare che tutte le valutazioni fatte negli ultimi anni dagli enti che esprimevano parere sulle manovre non hanno mai centrato l'obiettivo. In merito al superamento della cosiddetta legge Fornero, vorrei ricordare ai senatori presenti che le stime per i posti di lavoro generate da Impresa 4.0 per l'Italia prevedono una perdita di 200.000 posti di lavoro, controbilanciata da 200.000 posti di lavoro nuovi, con nuove competenze; quindi saldo zero, ma competenze e necessità diverse. Anche e solo per questo si dovrebbe essere positivi su questa misura. Quando si parla di blocco degli investimenti, vorrei ricordare che invece nella NADEF si parla proprio di voler sbloccare quegli investimenti che non sono stati compiuti nel passato e quando si fa riferimento al fatto che il Ministro delle infrastrutture stia di fatto bloccando gli investimenti, vorrei ricordare, in primo luogo, che a breve il Ministro riceverà un *dossier* sull'analisi che aveva richiesto sulle opere, in modo da definire su quali procedere e in che tempi; in secondo luogo, visto quanto scoperto dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, e cioè gli elevati profitti assicurati al concessionario, ritengo che il Ministro stia facendo bene, per interesse di tutti gli italiani, a verificare che cose simili non accadano in altri ambiti per opere seguite dal suo Ministero. Se è vero, come ha detto il collega Battistoni, che di buone intenzioni è lastricata la strada per l'inferno, vorrei dire che questa strada la stiamo purtroppo ormai percorrendo da tempo. È ora di costruire una nuova strada e se il 4 marzo è stata posta la prima pietra, questa NADEF è la via della costruzione di un nuovo percorso per l'Italia. Quando il senatore D'Arienzo, senatore dell'attuale opposizione che ha governato il Paese nell'ultimo quinquennio, ci accusa non aver messo un euro in più in aggiunta a quanto già stanziato su investimenti, ma di usare quelli del precedente Governo, Governo, prima di fare questa affermazione si è chiesto perché il Governo precedente non è stato in grado di spenderli? Egli ha involontariamente certificato che il Governo del Partito democratico non è stato in grado di effettuare gli investimenti per cui aveva stanziato risorse. Credo che il senatore Romeo abbia efficacemente risposto a questo punto. questo punto. La senatrice Bonino, che mi spiace non sia presente, ha detto che non c'è un profumo di investimento - solo lo 0,2 per cento - e che tutto o quasi è finanziato con il debito e quindi la soluzione sarebbe fare tutti investimenti; ma nel frattempo che partono investimenti, la gente che dovrebbe lavorare e vivere, deve arrancare? Siamo uno dei pochissimi paesi d'Europa a non avere uno strumento come il reddito cittadinanza. Sbagliano tutti gli altri Paesi o hanno sbagliato coloro che ci hanno governato finora? Senatore Manca, la questione del moltiplicatore è dibattuta fra UPB e il ministro Tria, vedremo nel tempo chi avrà ragione. Nel frattempo, però, vorrei farle presente che il moltiplicatore per il reddito di cittadinanza è alto in quanto è vero che si tratta di trasferimenti a famiglie ma sono famiglie tecnicamente con alta propensione al consumo, e traduco per chi ci ascolta da casa: sono famiglie che non avendo praticamente nulla non hanno propensione al risparmio e spenderanno i soldi ricevuti per i beni necessari per vivere, pertanto quei soldi torneranno immediatamente - e tutti - nel circuito, alimentando un circolo virtuoso di domanda-reddito-occupazione. In conclusione, ritengo comprensibili le preoccupazioni dei colleghi: comprensibili ma non condivisibili. Noi tutti, tutti, tutti, siamo stati scelti dagli italiani per cambiare le sorti del Paese ed è giunto il momento di farlo con una manovra che ci permetterà di recuperare la competitività e la posizione che l'Italia si merita in Europa e nel mondo.

una sola risposta puntuale al senatore Durnwalder in merito al tema delle autonomie. Il tema delle autonomie non è trattato perché la novità è che non si vuole trattare tale tema, nel senso che non si vuole incidere sull'autonomia delle Regioni Regioni a Statuto speciale, tant'è che si vuole estendere l'autonomia procedendo nell'autonomia differenziata su un percorso che è già stato avviato in alcune realtà. Al netto di questa precisazione puntuale, do alcune risposte ad una serie di questioni che sono state poste da diversi senatori e senatrici. Il punto chiave è la crescita, il PIL. Come mai siamo puntualmente ventisettesimi su 27? Negli ultimi anni siamo sempre ultimi, ventisettesimi su 27. In dieci anni abbiamo perso il 4,2 per cento mentre la media europea è +5,8, quindi 10 punti persi in dieci anni rispetto alla media europea. Come mai? La domanda ha una risposta complessa e rientra in alcune delle misure principali che sono state proposte nella Nota di aggiornamento che poi diventeranno oggetto di un testo puntuale nella legge di bilancio. Il primo tema che affrontiamo è quello del reddito di cittadinanza, tanto controverso però necessario. Il fatto stesso che già si era pensato di iniziare a introdurre qualcosa che andasse nella direzione di sostenere il reddito delle famiglie più in difficoltà fa capire che il problema c'è: il numero dei poveri in Italia è esploso dal 2012 in poi, questo è un dato di fatto, e quindi è opportuno affrontare il tema. Ma c'è l'altra metà della luna che riguarda le politiche attive del lavoro. Oggi noi abbiamo un sistema dei centri per l'impiego che sostanzialmente è un centro per l'impiego di chi lavora nel centro per l'impiego. *(Applausi dai Ma nel fare qualcosa andiamo anche a vedere ciò che già esiste. Io ho presente la realtà lombarda perché vengo da lì, negli ultimi cinque anni ero lì. In Lombardia, ogni anno, si avviano al lavoro oltre 100.000 giovani. Migliorabile anche questo dato, però sono oltre 100.000 giovani avviati al lavoro. Si dirà che quella è la Regione Lombardia. Perfetto, però abbiamo Regioni dove siamo a zero: da 100.000 a zero è evidente che qualcosa si può e si deve fare. Quindi, intervenire per rimettere in pista un sistema di politiche attive del lavoro serio che porti i nostri giovani a trovare un'attività è sacrosanto e doveroso. Questo è un punto fondamentale, un aspetto che crea sviluppo e crescita. Si tratta di un tema incontrovertibile. Per inciso, al senatore Patriarca che chiedeva delle cifre sui fondi sociali, faccio presente che la somma totale dei fondi sociali previsti vale circa 1,3-1,4 miliardi

Siccome non siamo i responsabili, ci stiamo attivando e penso che proprio nei prossimi giorni si troverà una soluzione per azzerare questi tagli, quindi dare la possibilità di andare avanti. avanti. Ricordiamoci, però, che ad oggi sono stati azzerati imponendo un taglio ben superiore al totale dei trasferimenti delle Regioni.

non si spende? Perché la spesa di investimento è stata bloccata, motivo per cui siamo al ventisettesimo posto su 27? Ci sono diverse questioni di carattere contabile, di carattere organizzativo,

Direte: sì, ma a fronte di una sentenza della Corte costituzionale che ha modificato una legge. Certo, una legge che noi orgogliosamente non avevamo votato perché sapevamo che era sbagliata. Quindi la circolare va a risolvere un errore fatto, purtroppo, e dico purtroppo perché questo negli anni ha bloccato tanti piccoli investimenti. E chi fa gli investimenti diretti sul territorio? Gli enti territoriali, i Comuni e le tanto bistrattate Province. Ebbene, con una circolare gli avanzi sono a posto. Tutto qui? No, ci sono tanti altri temi che dovremo affrontare: il fondo crediti di dubbia esigibilità, per esempio. Per inciso, la pace fiscale va a risolvere anche un pezzo di questo perché pulisce buona parte dei bilanci dei Comuni che sono bloccati da arretrati che non entreranno mai. *(Applausi dai chi fa materialmente gli appalti e perché non si fanno gli appalti di lavori pubblici? Non si fanno gli appalti perché noi riusciamo anche a complicare e a peggiorare le direttive europee, che già di loro non sono sempre una buona notizia. il codice degli appalti siamo riusciti a fare un capolavoro mettendo in piedi un sistema per cui per il progettista si fa la gara e ci vogliono sei mesi, poi si fa la gara per la ditta e ci vogliono altri sei mesi; sempre che non ci sia un ricorso e che l'ente

accelerarli. Nella Nota di aggiornamento e nella manovra che si fa viene prevista una misura importantissima, ossia la riduzione dell'IRES di nove punti, dal 24 al 15

bassa: un cambiamento radicale. In cambio cosa chiediamo alle imprese, a fronte di tale grande taglio di nove punti? Di investire e assumere, ossia di fare quello che serve per lo sviluppo del Paese.

Vi sono tanti impegni e tanti buoni propositi difficilmente non condivisibili: le risorse per la sicurezza, le nuove assunzioni per le Forze dell'ordine, gli investimenti nella giustizia, l'abbassamento della pressione fiscale, le risorse per il sociale e quelle per le pensioni. Tutto bellissimo, se non fosse che una cosa sono i desideri e un'altra è la realtà, perché purtroppo tutti sappiamo che non ci sono le risorse per gran parte delle vostre proposte e la soluzione non può essere quella di aumentare le spese di un Paese già oberato dai debiti. La vostra teoria del *deficit spending* e dell'impulso alla domanda interna non funzionerà se non sarà prima risolta una serie di altre problematiche. Serviva e serve, allora, un piano per la semplificazione burocratica, serve una giustizia più veloce, serve migliorare la produttività delle aziende a parità di costi, serve un piano per favorire gli investimenti privati, servono misure per abbattere il costo del lavoro a tempo indeterminato. è davvero un Governo di legislatura, che quindi guarda oltre le elezioni europee, in questa fase bisognava mettere al centro misure volte a modernizzare il sistema e a superare i *gap* strutturali rispetto al tessuto imprenditoriale e produttivo delle altre economie avanzate, che sono poi le ragioni fondanti della bassa crescita dell'Italia. Qui invece si fa una distribuzione di risorse attraverso nuovo debito, secondo la teoria che così crescerà il PIL. Le vostre previsioni sono inadeguate ed è inutile deridere professori di economia e ragionieri dello Stato o dire che dello *spread* non vi importa nulla. Questo vostro modo di fare e di comunicare non crea fiducia, ma contribuisce a destabilizzare e l'insicurezza delle persone è il più grande disincentivo a spendere, consumare e investire. L'insicurezza crescerà quando si accorgeranno che le misure che state raccontando non corrispondono alla realtà dei fatti, perché la chiamate *flat tax*, ma in verità è un innalzamento dei tetti di fatturato per le partite IVA con il regime forfettario. Lo chiamate reddito di cittadinanza, ma è un sussidio per l'accesso a beni di prima necessità per alcune specifiche e ridotte categorie di persone in difficoltà. Questo sussidio non è nulla di spettacolare e già esiste nella gran parte degli Stati europei e in Sud Tirolo. In quei Paesi il sussidio esiste senza che lo Stato decida cosa i cittadini possono comprare e cosa no. Poi la minaccia di sei anni di carcere è davvero una proposta assurda. Volete davvero introdurre un nuovo reato sull'uso immorale del sussidio? Ha ragione la collega Bellanova quando parla di «condono per i ricchi e carcere per i poveri». La chiamate pace fiscale, come a voler dire che è in corso una guerra tra i cittadini e l'erario, ma sarebbe meglio definirla una vittoria dei più furbi sulla pelle degli onesti, di chi paga le tasse e rispetta le regole, anche a costo di grandi sacrifici. Lo dico soprattutto ai Cinque Stelle, che dell'onestà hanno fatto la ragione fondante del loro impegno politico. Mettiamoci nei panni di un commerciante che ha sempre pagato tutto e che sa che il suo concorrente se l'è cavata con un salvacondotto. Mi dite che significato avrà per lui da oggi la parola onestà? Ci chiediamo, poi, cosa significhi attivazione della cosiddetta clausola di spesa, nel caso di una crescita che non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati. Quali spese verrebbero tagliate? Quelle in conto capitale o la spesa corrente? Quindi le misure che introducete potrebbero essere revocate? Chi oggi beneficia della quota 100 potrebbe essere richiamato al lavoro? Insomma, mi sembra tutto molto vago. Peraltro, rispetto al passato recente, ci muoviamo in un quadro più difficile: l'innalzamento delle barriere commerciali, la fine delle misure di sostegno della BCE, le incognite legate alla stabilità politica internazionale. In un simile contesto una manovra in disavanzo diventa ancora più rischiosa e una manovra al 2,4 per cento assume i contorni dell'azzardo. È un azzardo e non serve a nulla chiedere l'aiuto agli italiani, se nel frattempo i milioni di investitori che compongono il mercato stanno stanno già dicendo che del nostro debito non si fidano. Insomma, non credo proprio che i mercati vorranno bene all'Italia, come ha detto il vice presidente Di Maio. Così come non servirà a nulla continuare a prendersela con l'Europa, con i vari organismi nazionali e internazionali, che stanno solamente dicendo al Paese di non vanificare i sacrifici fatti in tutti questi anni per uscire dalla crisi. Perché, alla fine, pagheranno ancora una volta le giovani generazioni e i ceti meno abbienti. Quando si deve passare ai fatti, il Governo del cambiamento non è poi così abile come con le parole. La incredibile gestione dell'emergenza di Genova è sotto gli occhi di tutti. E quindi, altro che cancellazione della povertà, ma una manovra scritta con la penna dell'immediato tornaconto elettorale. Per questo, signor Presidente, dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo.

noi di Liberi e Uguali non possiamo certamente essere annoverati tra le vestali e i custodi dei parametri

percorsi, proposte che mettessero in discussione il *fiscal compact* e quegli stessi parametri. Quindi, tolta la retorica e tutte le frasi a effetto che si sono sentite in questi giorni nella discussione sulla Nota di aggiornamento, penso che dobbiamo andare alla sostanza di questa manovra. Questa certamente poteva essere una Nota di aggiornamento e anche di cambiamento radicale, ma - ve lo dico ancora una volta - pensate davvero che sia così? Le politiche di *austerity* e recessive hanno provocato vent'anni di stagnazione, in particolare in Italia

e peggiorare le proprie condizioni di vita, mentre il 20 per cento più ricco ha visto migliorare la propria situazione; sono quelle politiche che ci hanno spiegato che erano giuste le privatizzazioni, i tagli alla spesa sociale e alla previdenza, la flessibilità

alle pensioni minime a 780 euro e al reddito di cittadinanza. Per quanto ci riguarda, stiamo stati tra i primi in quest'Aula, anche nella scorsa legislatura, a presentare un disegno di legge sul reddito minimo garantito come misura di stampo universalistico. Tuttavia, anche in

qual è il contraltare a queste misure? Come sono - negativamente a nostro avviso - compensate? Sul piano fiscale ci si muove del tutto in linea con l'impianto di quelle

un'iniezione fortissima di politiche di progressività per superare l'elemento di ingiustizia nel sistema fiscale. E invece parlate di pace fiscale e di condono: questa sarebbe la novità?

tratta esattamente del contrario di un riorientamento del sistema fiscale verso una maggiore progressività. Aggredire la questione delle disuguaglianze e trovare le risorse significava avere il coraggio di mettere mano alla tassazione dei grandi patrimoni, ma di questo

In più, serve un'altra cosa per sostenere, anche in Europa, lo star fuori dai parametri, perché per sostenere il confronto con le istituzioni europee e l'ideologia deflazionista dei gruppi dirigenti europei

hanno la stessa idea di stampo neoliberista, quindi questo non garantirà affatto che si potrà cambiare il paradigma.

alle alleanze, quando si affronta uno scontro, ad esempio, con tutti i Paesi che più hanno sofferto quelle politiche di rigore. Torniamo sugli investimenti pubblici: lo 0,2

allargando le fasce della trattativa privata e degli affidamenti diretti, in pochissimi mesi? Veramente non so se vi illudete o volete illudere. Come vedete, le questioni

ci saremmo augurati il cambiamento radicale, proprio per mettere in discussione - perché siamo coscienti di quello che è accaduto a causa delle politiche di rigore, di *austerity*, in tutta l'area dell'eurozona, a parte alcuni pochi Paesi, come la Germania - quello che è accaduto, le conseguenze sulla vita dei cittadini e e l'aumento della povertà e delle disuguaglianze. Ma tutto questo purtroppo - ahimè - non c'è, e le cose buone e condivisibili sono immediatamente contraddette da altre misure che sono di stampo assolutamente regressivo. Per tutti questi motivi, i senatori di Liberi la Nota di aggiornamento, ma ci asterremo invece sulla risoluzione per quanto riguarda lo scostamento. Ci asterremo perché noi siamo per superare i parametri e vi sfidiamo su questo, tant'è, signor Presidente, che annunciamo che oggi stesso noi presenteremo un disegno di legge costituzionale per rivedere il pareggio di bilancio in Costituzione; e vedremo se saprete davvero accettare la sfida, sfida, non solo a parole e con gli *slogan*, ed arrivare ad un orizzonte diverso, che metta in discussione il *fiscal compact* e le politiche di rigore che ci hanno imprigionato in tutti questi anni.

noi non siamo spaventati dal fatto che il Governo abbia scelto di fissare al 2,4 per cento il rapporto *deficit*-PIL: tutto sommato, preferiamo un Governo che lo dichiari sin dall'inizio, nel preventivo, e mantenga questo impegno, rispetto ai Governi che invece fissavano alla metà, all'1-1,5 per cento il rapporto *deficit*-PIL nel proprio preventivo, a consuntivo si ritrovavano con le stesse cifre e adesso hanno pure il coraggio di fare la predica agli altri. E non siamo spaventati nemmeno dallo *spread* sopra 300 di queste ore: conosciamo queste dinamiche. Noi abbiamo vissuto le stagioni di un Governo legittimo, l'ultimo Governo legittimo eletto dai cittadini, perché dal Governo Monti in

quel Governo venne spazzato via da uno *spread* a 600, dopo che per un anno ha combattuto con valori sopra quota 400: figuratevi che paura ci può fare quota 300! Peraltro, sono altre le forze politiche che, quando l'Italia è sotto attacco, fanno il tifo per il nemico pur di andare contro il Governo del proprio Paese se stanno all'opposizione. Noi no. Noi non apparteniamo a questa genia, siamo troppo italiani per volere il male della nostra nazione. E non ci impressiona neanche più di tanto che la Banca d'Italia, la Corte dei conti, il Fondo monetario, le agenzie di *rating*, l'Ufficio parlamentare del bilancio, l'Istituto nazionale di statistica abbiano tutti (dico tutti, e ne risparmio molti) bocciato le previsioni di crescita economica che il Governo sostiene di poter raggiungere per rendere sostenibili questi nuovi debiti. Governo che, oltretutto, per bocca del ministro Tria dichiara, anche con molta prosopopea, di aver fatto persino stime prudenti, addirittura pessimistiche, quindi che cresceranno più di quanto scrivono, se le cose andranno davvero come pensano e come dicono. Quello che ci spaventa davvero in questo quadro è l'atteggiamento di superficialità,

messo in campo per affermare i diritti e bisogni del popolo italiano, avendo però le spalle larghe per reggere l'urto e le idee giuste per sfidare il sistema e il pensiero dominante, o si tratta, invece, di irresponsabilità?

vincerla? Non è poi un grande gesto patriottico, e nemmeno una politica particolarmente popolare trascinare l'intera nazione in un'avventura che può avere come risultato, non la conquista di maggiore ricchezza, benessere e felicità, ma, all'opposto, rischia di aprire una nuova drammatica stagione, che può aprire le porte alla speculazione finanziaria, fino ad arrivare di nuovo allo spettro della *troika* e del commissariamento sostanziale dell'Italia. A noi non manca il coraggio di accettare una sfida impegnativa e vorremmo incontrare sul nostro percorso compagni di strada capaci di condividere la bellezza di una sfida esaltante. Per questo vogliamo mettere in guardia il Governo, perché sta porgendo il collo alle zanne della speculazione, speculazione che, notoriamente, non ha pietà ed è pronta ad affondare nella carne viva per realizzare i propri disegni. Si mostra, infatti, il collo alle zanne della speculazione finanziaria quando si sceglie di destinare alla spesa corrente gran parte del nuovo debito previsto di distribuire reddito e pensioni di cittadinanza pensando che questa pioggerellina di assegni di sussistenza possa far ripartire davvero l'economia reale e i consumi. Ci si espone quando si racconta, come ha fatto il ministro Tria, che l'unica politica per il Sud presentata dal Governo è il reddito di cittadinanza e non il lavoro, lo sviluppo e le infrastrutture. Non ci sorprende, d'altronde, che un Governo composto da una forza con un'origine, un radicamento e una cultura marcatamente settentrionale, se non addirittura nordista, non abbia la necessaria attenzione e sensibilità verso il Mezzogiorno d'Italia e conoscevamo la debolezza culturale della proposta economica grillina, fondata sull'assistenzialismo e sulla logica del sussidio di stato. Il risultato non poteva che essere questo, abbandonando il Sud a un destino di sottosviluppo. Si resta perplessi quando, da un lato, assistiamo al conflitto aperto e irrituale tra i capi del Governo e il presidente dell'INPS, colpevole di difendere l'assetto pensionistico della riforma Fornero, e, dall'altro, lo stesso Governo dichiara nel DEF (andate a leggere a pagina 73 quello che scrivete voi, che scrive questo Governo) che la riforma Fornero ha garantito una maggiore equità tra le generazioni, avendo migliorato in modo significativo la sostenibilità grazie a requisiti di accesso più elevati per le pensioni di vecchiaia. Ci chiediamo qual è la linea del Governo: «Fornero infame», come si grida nelle piazze, o «Lode a Fornero», come si legge nei vostri documenti economici? Al di là delle polemiche, sulle pensioni come su tanti altri aspetti, naturalmente attendiamo la legge di bilancio per fare una vera discussione di merito e portare le nostre proposte, cui discuteremo. Prima tra tutte, noi riteniamo sia una vera priorità raddoppiare le pensioni di invalidità, perché la vera priorità non è portare le pensioni minime di chi non ha versato contributi

fisica o psichica e che oggi è costretto a vivere in maniera miserabile con 200, 300, quando va bene 400 euro di pensione e sperare solo nell'aiuto e nel conforto dei propri cari. Questa è la vera emergenza e spero che non il Governo, né l'opposizione, ma tutto il Parlamento voglia su questa questione mettere la parola fine e dare una risposta giusta e sacrosanta a chi ne ha davvero bisogno. bisogno. Se volete combattere davvero una guerra giusta e sperare di invertire il *trend* della crescita, quel *trend* che vede l'Italia sempre in coda quando le altre nazioni crescono e sempre prima in decrescita in tempo di crisi, e di riuscire a farlo, oltretutto, mentre tutte le previsioni macroeconomiche descrivono un mondo che rallenta o che rischia una nuova crisi, tra dazi, guerre commerciali, prezzo del petrolio in crescita, crisi e conflitti mediorientali e di altre aree di conflitto, bolle speculative pronte ad esplodere ciclicamente, dovete cambiare la politica economica che ci state proponendo. Spostate i 10 miliardi che butterete nel reddito di cittadinanza o almeno una parte, che nemmeno riuscirete a spendere nel corso del 2019, in attesa di riformare i centri per l'impiego, approvare leggi e circolari, esaminare milioni di domande, organizzare i corsi di formazione le attività - perché l'avete promesso voi che non resteranno sul divano, questi 6 milioni di persone, ma andranno a fare lavori socialmente utili o corsi di formazione - che non inizieranno il 1° gennaio. Spostate questi soldi verso le politiche fiscali e gli investimenti, abbiate il coraggio - almeno voi della Lega, che con noi avete condiviso questo programma economico e di Governo - di abbattere da subito il prelievo fiscale sulle famiglie e sulle imprese, non solo sulle imprese. La misura che avete proposto per le piccole e medie imprese è, come si dice qui, una romanella che non cambia la classifica. La pressione fiscale prevista nel vostro DEF (perché una volta che fate la Nota di aggiornamento diventa il vostro documento programmatico) resta drammaticamente e clamorosamente ancorata al 42 per cento, altro che *flat tax* al 15 per cento! Misure come quella dell'abbattimento fiscale, entrano subito in vigore: dalla busta paga di gennaio, mettono i soldi nelle tasche dei cittadini, che avranno così maggiore propensione alla spesa e ai consumi, di imprenditori che assumeranno di più perché produrranno di più e gli costerà di meno farlo. Questa è la vera crescita che serve. del Governo giallo-verde venite spesso sfottuti dai pensatori del pensiero economico classico perché siete ritenuti i sostenitori della decrescita felice, una critica che molti vi rivolgono senza aver mai nemmeno letto una riga di Serge Latouche. Il problema vero è che se non raddrizzate la rotta all'Italia non spetterà una stagione di decrescita felice (magari, almeno sarebbe felice e consapevolmente cercata) ma una tristissima stagione di decrescita infelice. È per questa ragione e per quelle illustrate nella proposta di risoluzione a firma di tutti i senatori del nostro Gruppo che Fratelli d'Italia voterà contro la Nota di aggiornamento al DEF. Signor Presidente, onorevoli senatori e onorevoli senatrici, la Nota di aggiornamento del Governo non sta in piedi, è scritta sulla sabbia. La Lega e il MoVimento 5 Stelle ci raccontano la fiaba di Bengodi: più investimenti, più crescita, tutti in pensione cinque anni prima, reddito e pensione di cittadinanza per 6 milioni di persone. La realtà è completamente diversa, è la realtà di una manovra sbagliata e pericolosa, che rischia di portarci fuori strada. Ci avete presentato delle previsioni inattendibili che sono state bocciate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e criticate dalla Banca d'Italia, dall'ISTAT e dalla Corte dei conti. La reazione della maggioranza, la vostra reazione, è stata all'insegna della delegittimazione e degli attacchi personali di fronte a queste critiche. I professoroni dell'Ufficio parlamentare di bilancio la Banca d'Italia che farebbe meglio a presentarsi alle elezioni, il presidente dell'INPS che deve dimettersi e, persino, come avete scritto nella vostra risoluzione, l'azzeramento del Fondo per il pluralismo dell'editoria, perché i giornali scomodi è meglio che chiudano. *(Applausi dal Gruppo PD)*. della libertà nel nostro Paese. Sono attacchi inaccettabili, signor Presidente, perché rivolti contro autorità indipendenti e contro la libera stampa, contro chi ha la sola colpa di tenere la schiena dritta nei confronti di chi comanda. Voi avete presentato una relazione ridicola al Parlamento, che non contiene alcun piano di rientro, come richiederebbe la Costituzione e la legge di contabilità. Con l'Europa siete ai ferri corti.

Questi proclami, che ci riportano indietro di ottant'anni di balcone in balcone, non hanno portato bene né al Paese, né a chi ha pronunciato quelle parole. E chi oggi pensa di difendere l'Italia, andando a testa bassa contro tutto e contro tutti, non ci porta da nessuna parte, fa solo del male agli italiani, a partire da quelli che hanno votato i partiti dell'attuale maggioranza. la manovra triennale è coperta per il 70 per cento da *deficit.* Il *deficit* non è un tabù di per sé, dipende se è sostenibile e da come viene utilizzato. Le manovre dei Governi Renzi e Gentiloni Silveri sono state espansive e hanno aiutato l'Italia ad uscire dalla recessione, a creare posti di lavoro e rimettersi in piedi.

Nel 2021, al termine del triennio, il debito pubblico sarà più alto di 110 miliardi di quello che avremo a fine del 2018: 110 miliardi caricati sulle generazioni future, 110 miliardi di debito in più che mettono a rischio i risparmi delle famiglie italiane. È un film già visto negli anni Ottanta, che non ha un lieto fine, cari colleghi, perché il conto di quel film lo stiamo pagando ancora oggi e dovremmo evitare di ripetere gli errori del passato. Vi proclamate il Governo del cambiamento, avete parlato anche in quest'Aula di discontinuità, di Terza Repubblica, ma qui di essa non c'è traccia: stiamo tornando nella peggiore stagione della Prima Repubblica del Paese. Tutto questo *deficit*, secondo quello che scrivete, dovrebbe servire a riattivare la crescita ma, in realtà, va quasi tutto nella parte corrente: lo *stop* all'aumento dell'IVA che, peraltro, si ferma nel 2019; quota 100 per le pensioni e non si capisce se sia temporanea, come detto dal ministro Tria o permanente; il reddito di cittadinanza che parte con buone intenzioni e rischia di replicare il peggiore assistenzialismo di Stato. sono gli investimenti, naturalmente, di cui ha parlato anche il sottosegretario Garavaglia. Peccato che rimangano le briciole per gli investimenti, perché le risorse per gli investimenti sono meno del 15 per cento della manovra triennale. Per il resto: tagli alla scuola, zero per l'università, zero per la ricerca, zero per il Mezzogiorno e nulla per il futuro di questo Paese. Ha ragione lo storico Emanuele Felice che ha scritto che così firmiamo il nostro declino, perché in questa manovra non c'è futuro per il Paese ma c'è solo il declino, la decrescita, tutto tranne che la decrescita felice. il ministro Tria ha insistito molto sugli investimenti in Commissione. Ha ragione, perché vanno rilanciati, però dovrebbe mettersi d'accordo il ministro Tria con il ministro Toninelli perché mentre la mano destra - Tria - dice che gli investimenti li vuole rilanciare, la mano sinistra - Toninelli - non ha ancora sbloccato i 36 miliardi stanziati stanziati dal Governo Gentiloni Silveri, ha bloccato grandi opere per 19 miliardi e ha tolto i soldi alle periferie, cioè alla parte del Paese che andrebbe sostenuta e dove prioritariamente bisognerebbe investire. Infine, mi avvio alla conclusione: la pace fiscale. Cari amici del Movimento 5 Stelle, pace fiscale? È la fiera dell'ipocrisia. Abbiate il coraggio di chiamare quella misura con il suo vero nome: è un condono! È uno schiaffo per i contribuenti onesti, per chi le tasse le paga fino all'ultimo euro ed è un favore per chi le tasse non le ha mai pagate e continuerà ad evaderle. Ho finito, signor Presidente. Questa manovra ci porterà fuori strada. Ci appelliamo al Governo e alla maggioranza: tornate nel mondo reale. Nel 2019 dovremo collocare 400 miliardi di euro di titoli di Stato. Voi avete bisogno di un capro espiatorio, continuamente, è questa la narrazione dei sovranisti, ma il problema di questo Paese non è l'Europa, sono i risparmiatori, che dobbiamo convincere giorno dopo giorno a comprare questi titoli di Stato. Lo *spread* era 130 prima delle elezioni, oggi è sopra quota 300 e le tabelle della vostra Nota ci dicono che già quest'anno pagheremo due miliardi in più di interessi, 11 miliardi in più nel triennio 2019-2021 che diventano 18 miliardi in più di interessi con la vostra manovra. Questo è il prezzo della vostra confusione, delle vostre contraddizioni, della vostra demagogia e quelli sono soldi dei contribuenti, bruciati sull'altare della demagogia, tolti ai servizi pubblici, tolti agli investimenti e tolti alla riduzione della pressione fiscale. Cambiate strada, cambiate questa manovra, piantatela di giocare con i soldi dei cittadini. Pensate un po' meno alle prossime elezioni europee e un po' di più al futuro di questo Paese e al futuro dei nostri giovani e fatelo subito, prima che sia troppo tardi.

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà un breve intervento tecnico che però si riaggancia al concetto espresso, con una certa concitazione in questo momento, dai banchi dell'opposizione, cioè la giusta esigenza di evitare gli errori del passato. Vi parlerò di qualche numero, anzi di percentuali: 40,9, 5,7, 31,9 e 6,7. Cosa sono queste percentuali? il riassunto della parabola politica dei due estensori della cortese lettera che il 5 ottobre scorso è stata ricevuta dal nostro Governo, una parabola politica sulla quale domando la vostra riflessione costruttiva. 40,9 è quella che fu raggiunta dal Partito Socialista francese al secondo turno delle legislative del 2012; Pierre Moscovici divenne Ministro dell'economia e delle finanze e, visto che ci interessano tanto le percentuali, dal 2012 al 2014 mantenne quella carica, facendo in media il 4,3 per cento di *deficit*. Poi andò a fare il Commissario per gli affari economici dell'Unione europea ma due anni dopo, nel 2016, il *deficit* francese è ancora al 3,4 Qualche giornalista, in qualche conferenza stampa, chiese a Jean-Claude Juncker come mai le cose andassero così e bisogna ricordare la risposta di Juncker quando si accusano i Ministri del nostro Governo di non mostrare sufficiente spirito europeista. Bisogna ricordare che Juncker rispose che la Francia fa il 3,4 e lo può fare perché è la Francia. Queste parole, legittimando l'idea che esistano figli e figliastri, fanno molto più male al progetto europeo di qualsiasi giusta rivendicazione del nostro Governo. *(Applausi Ma ci vengono date pillole di fondamentali macroeconomici: ci viene detto che però loro hanno meno debito pubblico. Ha fatto benissimo il nostro Capogruppo, prima, a ricordare che il debito pubblico non è l'unico elemento di giudizio di un sistema economico: esiste, per esempio, anche il debito estero. Parliamo del debito pubblico: dal 2007 al 2018 quello francese è aumentato di 32 punti; quello italiano di soli 30. Parliamo del debito estero: la posizione debitoria netta francese è peggiorata di circa 20 punti e la nostra è migliorata di circa 20 punti, nello stesso lasso di tempo. Quindi - come dire? - non riporrei troppe speranze nel fatto che la Francia possa restare un esempio virtuoso a lungo. Vi parlo adesso del 31,9 - avrete capito dove voglio andare a - ovvero la percentuale che il partito lettone Unità raggiunse alle politiche del 2010 (primo ministro Valdis Dombrovskis, eletto un anno prima, nel 2009). alle ultime elezioni questo partito ha ottenuto il 6,7. Come spieghiamo questo tonfo? Non essendo Dombrovskis la Francia, non poteva permettersi di non fare austerità; l'ha fatta e qui arriva subito il Pierino della macroeconomia, che fa notare che comunque in Lettonia la disoccupazione è scesa dal 19 all'11 per cento. D'accordo, allora vi spiego anche come è successo: la diminuzione c'è stata perché in un Paese che riceve circa il due per cento del suo PIL di sussidi dall'Unione europea, il 10 per cento della popolazione in età lavorativa è emigrata; ha esportato quindi lavoratori - e anche tensioni macroeconomiche - in altri Paesi. Questo lo dico *pro veritate,* non con spirito di rivalsa, ma per riflettere su qual è il modello al quale ci viene chiesto di conformarci. Dovremmo ricordarci tutti che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio, e i due firmatari della lettera al ministro Tria a casa loro il cattivo esempio non lo potranno dare più. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Questo solo per dire che se noi siamo barbari, come si chiama il «Financial Times», che ringraziamo per la sua attenzione, non è perché in Italia ci sia stata un'epidemia di populismo, è solo perché la democrazia

perché in tutta evidenza ha aumentato la conflittualità sociale e anche quella internazionale in Europa, e lo ha fatto perché viziato da un'ipocrisia di fondo, dalla quale dovremmo finalmente liberarci: quella che consente di spacciare come scelte tecniche quelle che in fondo sono decisioni politiche,

queste regole sono state applicate ai nemici e interpretate o riscritte per gli amici, come quando la Germania violò - cosa che il collega Renzi ha ricordato in altri tempi - la regola del tre per cento e questa regola venne subito corroborata corroborata con una serie di scappatoie, del tipo: i tedeschi, però, hanno fatto le riforme, quindi possono fare come gli pare. Ci accusate di aver scritto un libro dei sogni, ma poi vi inchinate di fronte a un feticcio totalmente arbitrario e contestato da una parte della comunità scientifica che è il prodotto potenziale, cioè che cosa sarebbe il PIL, il sogno di un PIL, in un mondo in cui tutti lavorassero, cosa che però non possono fare perché viene impedita esattamente da quelle regole basate sul concetto di PIL potenziale e di *output gap*. Questo - se permettete - è un paradosso sgradevole. Fa bene quindi, anzi benissimo, il Ministro a ricordare, - cito testualmente - «la persistente debolezza delle condizioni cicliche» del nostro Paese «non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale».

Secondo noi, questo DEF è la manovra corretta da fare ora, in termini sia congiunturali che strutturali. Poco meno di quattro mesi fa vi ricordavo che il ciclo economico espansivo in corso negli Stati Uniti risultava essere il secondo più lungo nella storia del dopoguerra, e ieri abbiamo visto qualche scricchiolio; ricordavo anche le difficoltà nelle quali incorrevano alcuni nostri *partner* europei, e due giorni fa l'agenzia Reuters si stupiva del fatto che l'economia tedesca inanelli un crollo della produzione dietro l'altro. Non ci vuole molto a capire che un modello fallimentare non è un gioco a somma zero, ma un gioco a somma negativa, ed è per questo che chi è realmente animato da uno spirito di genuina, positiva e costruttiva fratellanza europea deve contestarlo. In queste condizioni, non possiamo più contare sul tiro della domanda estera, e dobbiamo essere pronti a contrastare gli effetti di *choc* finanziari che rischiano di arrivare dall'altra parte dell'Oceano o dai mercati emergenti. A questo scopo, occorre rilanciare la domanda interna ed è precisamente questa la filosofia del DEF, che viene messa in opera in primo luogo con le misure di sostegno dei redditi e degli investimenti e con l'alleggerimento della pressione fiscale. è soprattutto un gesto di disobbedienza civile: respingere manovre recessive nelle condizioni attuali ci aiuterà a promuovere un dibattito sul significato della nostra convivenza in Europa, esattamente come fermare una certa nave quest'estate - oltre a salvare un discreto quantitativo di vite umane, non più incentivate a mettersi a rischio - ha promosso un dibattito sulla comune gestione dei nostri confini e dei flussi migratori.

Per questo motivo, a questo programma, andrà il convinto voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito

Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto traggo le fila di una serie di considerazioni che sono state fatte dai colleghi Grazie a diversi aspetti di questa Nota di aggiornamento al DEF e naturalmente sono propedeutiche alla successiva manovra di bilancio, che è quello che tutti ci ci aspettiamo di vedere, prima o poi (perché per ora la sua diffusione è stata solo orale e tralaticia, attendiamo che prima o poi la carta o il supporto informatico compaiano e ci consentano di giudicare più approfonditamente di cosa si tratta). I numeri, però, ci sono già,

ci aspettavamo un respiro più ampio, una visione, un'idea di Paese e una rappresentazione di quel Governo del cambiamento attraverso atti spalmati sulle poste di bilancio dello Stato.

nell'avventatezza; quella parte in cui quelle che definite «sfide» sono da noi considerate un azzardo, un rischio; e vi spiego perché. Non sono qui per fare affermazioni apodittiche; ognuno di noi ha portato la sua motivazione e anche noi lo faremo. Ho apprezzato molto le considerazioni del senatore Marsilio che ha espresso con grande buon senso, molta obiettività e soprattutto con l'orgoglio della sua storia, che è anche la nostra storia e dell'ultimo Governo eletto dagli italiani nel 2008. Grazie

e giustamente il collega Marsilio ha detto: non saremo certo noi a iscriverci al partito di "forza *spread*"*.* Per carità, noi lo abbiamo subito lo *spread*, vergognosamente. siamo stati oggetto di un inganno dello *spread* che mai e poi mai potremmo rivoltare come argomento politico nei confronti dei nostri avversari, che per noi sono - lo ripeto - avversari e non nemici, che devono essere ascoltati e controdedotti, non delegittimati.

Noi sappiamo che il *deficit* non è altro che debito futuro che impatterà sulle spalle, sulla pelle e sulle tasche di tutti noi, di tutti gli italiani, ed è degli italiani che in questo momento ci dobbiamo preoccupare, perché siamo qui a rappresentarli. L'*extra* *deficit*, che sarà debito futuro, non è ‑ come tutti gli strumenti, buono o cattivo in se stesso; dipende da come lo si usa. È buono se lo si usa per fare investimenti prospettici

di questo Documento che doveva essere la grande visione del cambiamento di questo Governo a due teste: una ci piace, l'altra molto meno, ma sono due teste che non hanno idee particolarmente originali in questo Documento.

chiedo un prestito e lo uso per fare innovazione nella mia azienda (innovazione di prodotto, di processo e di percorso), arricchisco me stesso, la mia famiglia e i miei dipendenti; giovo ai miei fornitori e faccio circolare i consumi.

che contraggo nei confronti della banca a cui ho chiesto il prestito faccio speculazioni sbagliate, sbagliatissime, e quello che resta in un momento di follia me lo gioco alla *roulette*, allora non faccio debito sano, ma azzardo puro, che impoverirà me stessa e la mia famiglia. Credetemi che queste non sono considerazioni peregrine. Vedo il ministro Salvini

dal Gruppo FI-BP)*. Lo diremo agli italiani che non devono perdere la speranza, nel momento in cui - Dio non voglia, perché noi tifiamo Italia - quello che sta succedendo sui mercati impatterà sui loro risparmi, sui loro mutui, sui loro prestiti e sulle loro famiglie. Amici miei, lo ripeto ancora una volta: non sono, insieme al mio Gruppo, mai stata timida rispetto alle critiche verso quei burocrati e quei commissari che pretendono di farci la lezione e di insegnarci come dobbiamo governare e che spesso confondono il rigore dei conti pubblici con il *rigor mortis* dell'economia. Quelli non siamo noi. A noi va bene fare debito, a noi va bene investire su noi stessi, ma come? Abbassando le tasse sulle imprese, sulle famiglie e sugli italiani nel complesso; questo non avviene

poco più di 400.000 partite IVA che già si giovavano e ora si giovano di un regime semplificato rappresentino l'applicazione della *flat tax*. Cinque scaglioni: questo è un regime non semplificato, ma complicato, per l'1 per cento dei contribuenti. E il

L'unica cosa che veramente funziona non è il pannicello caldo di una finta riduzione fiscale per l'1 per cento dei contribuenti, ma è un grande *shock* fiscale per il Paese. Quello e solo quello può rappresentare quell'inversione di tendenza di cui il Paese ha bisogno. Attenzione a non trovarci in mano un grande libro dei sogni perduti: gli italiani non ce lo perdonerebbero.

una notizia tragica, ma che purtroppo non ci può stupire, perché purtroppo questo non è un Paese che abbia un atteggiamento

Il reddito di cittadinanza è un altro tema che si ricollega strettamente a quello di cui ho appena parlato, cioè fare debito per fare cose utili. Se si fa debito per fare azzardo, il debito si rivolterà contro di noi. Il reddito di cittadinanza, colleghi, intercetta il bisogno il bisogno di agevolare il percorso al lavoro e il bisogno di dare assistenza a chi non ce la fa. Il reddito di cittadinanza, così come è strutturato in questo provvedimento, che è molto nebuloso, ha la "felice" capacità di ottenere il peggio di entrambe le cose: disincentiva il lavoro e stabilizza la povertà. alimenta il lavoro nero e rischia di aumentare le truffe nei confronti dei cittadini onesti. Vogliamo soddisfare i bisogni delle persone che non ce la fanno da sole, ma non così. Ascoltate le nostre ricette, a cui rinvio e che sono contenute nel nostro documento, che avete cassato senza nemmeno discuterlo. Noi lo abbiamo discusso e continueremo, insisteremo, combatteremo e lotteremo, perché le nostre convinzioni, le nostre ricette di buon governo economico, di sviluppo economico e di sostegno delle famiglie e delle imprese insieme, possano prevalere su ricette depressive, che non corrispondono alla nostra filosofia economica. Signor Presidente, avete capito che il nostro voto sarà assolutamente contrario

In questo Documento è riassunto tutto il nostro sogno, il sogno sotto il quale Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio ci hanno raccolto e accolto sin dal lontano 2009 e ci hanno portato nelle istituzioni nel 2013.

bloccato da una burocrazia asfissiante e da politiche restrittive. Il nostro è un atto di grande coraggio, per ridare serenità ai cittadini italiani, che per troppi anni hanno vissuto una politica di lacrime e sangue, hanno dato molto e ricevuto poco. Le regole europee di austerità negli ultimi anni non hanno prodotto i risultati auspicati: questo è sotto gli occhi di tutti, non lo possiamo negare e voi non lo potete negare. Non solo i conti non sono rientrati nei parametri stabiliti dall'Unione europea, ma il benessere degli italiani è sensibilmente diminuito. A dimostrarlo è il tasso di disoccupazione, pari al 10 per cento circa, mentre quello giovanile raggiunge addirittura il 31 per cento (le vostre politiche europee). La crescita dell'economia reale La crescita dell'economia reale è tremendamente lenta e ben lontana dai livelli pre-crisi. Siamo un Paese stanco, che viaggia a una velocità totalmente diversa rispetto a quella degli altri Stati membri. La Nota di aggiornamento al DEF presentata dal nostro Governo ha suscitato numerose perplessità. Sinceramente non le comprendo. Siamo consapevoli del fatto che si tratta di una manovra audace, ma questo è il momento in cui o si ha il coraggio di operare con delle scelte radicali e decisive, come chiesto dal popolo con il voto del 4 marzo, o il grido dei nostri dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Per questo motivo sono convinta che non bisogna lasciarsi trasportare dall'onda emotivamente instabile dei mercati. Le nostre prospettive di crescita future sono chiare e prospere lo dimostreremo. Il Documento di economia e finanza, presentato ad aprile dal precedente Governo, sebbene contenesse le politiche economiche restrittive Le previsioni di crescita del PIL per il 2018 erano pari all'1,5 per cento, mentre ad oggi il livello di stima si attesta all'1,2 cento. Per non parlare dei dati tendenziali 2019-2020: cifre ben diverse da quelle presunte. Volevate far crescere il Paese senza investire; su questo non avevate delle perplessità. La nostra manovra - è vero - prevede per il 2019 un rapporto *deficit*-PIL del 2,4 per cento, in linea con quelle che il vecchio Governo utilizzava per i regali alle banche e agli amici. Oggi invece ci si chiede di ascoltare i mercati, perché avete troppe perplessità. Ecco, noi vogliamo ascoltare i cittadini e prevediamo la riduzione del rapporto debito-PIL, oggi al 131,2 dal Gruppo PD).* Sono queste le cifre che ci permetteranno di rispettare i vostri vincoli europei e, al contempo, di garantire una qualità di vita dal Gruppo PD).* Per evitare di incidere sulle tasche dei cittadini, sulle imprese e quindi sull'economia in generale, l'azione del Governo inizierà bloccando l'aumento dell'IVA, quell'aumento Non meno importanti sono le azioni rivolte a destinare risorse agli investimenti pubblici, leva fondamentale per la crescita del nostro Paese. È impegno del nostro Governo sostenere gli investimenti in un'ottica che consideri sempre il rapporto costi-benefici di ogni progetto, con opere innovative e sostenibili. Si tratterà di misure che andranno a migliorare il livello di qualità delle infrastrutture del nostro Paese, rendendolo sempre più competitivo e attrattivo per gli investimenti. Anche la pressione fiscale, oggi con una media del 42,2 per cento, subirà una riduzione con l'innalzamento delle soglie del regime semplificato per imprese, professionisti e artigiani. invece, si applicherà la riduzione della tassazione sugli utili reinvestiti in macchinari e nuove assunzioni. Vogliamo poi parlare degli interventi sulla giustizia, quelli che il precedente Governo del PD si è dimenticato di fare, come il DASPO ai corrotti? Ecco, noi l'abbiamo fatto. Siamo sicuri che in un Paese che finalmente è impostato sulla legalità tutti vorranno venire ad investire. Grazie all'introduzione a regime della fatturazione elettronica, alla riduzione degli adempimenti fiscali e all'abolizione del redditometro si attuerà quella semplificazione di cui tanto si parla e che libererà tempo prezioso ai nostri imprenditori. *(Commenti del Gruppo PD).* Non solo, questo ci aiuterà a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, piaga del nostro Paese, e riporterà in vita un sano rapporto tra fisco e contribuenti. Basta contribuenti e imprenditori oppressi dal fisco! I contribuenti che si sono visti portare via la propria abitazione perché in difficoltà economica; gli imprenditori che hanno dovuto scegliere tra pagare le tasse o i propri dipendenti a causa delle vostre leggi non dovranno più esistere.

nel ciclo economico del Paese. Oltre alla semplificazione e alla riduzione della pressione fiscale, il Governo agirà al fine di tutelare le imprese per rafforzare il il contesto in cui le imprese stesse operano. Ne sono esempio la tutela del *made in Italy*, la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, il rafforzamento del piano impresa 4.0, la promozione dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Inoltre, il Governo, come ha già dimostrato con il decreto dignità, è impegnato a migliorare l'inclusione sociale, a lottare l'inclusione sociale, a lottare contro il precariato e a incentivare l'occupazione giovanile. Al fine di raggiungere questi obiettivi, risulta imprescindibile il superamento della legge Fornero, che ha creato numerosi squilibri generazionali. L'attuale sistema previdenziale garantisce certamente la stabilità finanziaria nel lungo periodo, ma blocca il *turnover* delle risorse umane nel medio periodo. Per questo assistiamo a migliaia di giovani costretti a scappare

di andare finalmente in pensione e ai nostri giovani di poter entrare nel mondo del lavoro, costruirsi un futuro e, chissà, una famiglia. Come abbiamo sempre promesso, rimborseremo anche i risparmiatori truffati; risparmiatori truffati due volte: prima dalla mala gestione delle banche con la complicità di chi non ha voluto vedere o ha fatto finta di non vedere e poi dalla politica, dal vecchio Governo PD che in un giorno gli ha azzerato i risparmi senza battere ciglio. Ultimo, ma non ultimo, il reddito di cittadinanza, misura progettata per contrastare la povertà, rafforzare la coesione sociale e stimolare le politiche attive del lavoro. Il MoVimento 5 Stelle da sempre è impegnato a istituire questa misura anche in Italia, già presente in tutti i Paesi europei. Si tratta non solo di un investimento verso le componenti più vulnerabili per far sì che queste tornino a partecipare pienamente al progresso della società, ma anche uno strumento di stimolo alla domanda aggregata. Il MoVimento 5 Stelle è nato per essere vicino ai cittadini e pertanto voterà favorevolmente alla Nota di aggiornamento al DEF, per avere finalmente una manovra a favore della felicità degli italiani. State tranquilli. Sarà la fiducia dei cittadini in questo Governo a conquistare quella dei mercati. Alla faccia delle vostre perplessità!

all'azzeramento dei fondi per l'editoria ed il pluralismo, penso agli interventi sulla Avvocatura dello Stato, che sostanziano un'idea di Governo autoritaria. un nostro emendamento calibrato su obiettivi che dovrebbero essere condivisi da chiunque sia chiamato a responsabilità politiche e istituzionali nel Paese. velocemente i quattro punti su cui poggia la nostra proposta, attraverso interventi sostitutivi e non aggiuntivi a quelli proposti nella risoluzione di maggioranza e che esprimono una visione di politica economica reale, che guarda ad un'occupazione vera e al sostegno alle famiglie come contrasto alla povertà. Il primo chiaro impegno è la riduzione del costo del lavoro, non del numero dei lavoratori come con il "decreto disoccupazione". Per incrementare occupazione stabile è necessario andare a tagliare il cuneo contributivo, per i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, e noi proponiamo di farlo con un punto all'anno per i prossimi quattro anni. Il secondo è favorire la ripresa degli investimenti; durante gli anni di Governo di centrosinistra sono stati sbloccati circa quattro miliardi di avanzi e con la sentenza n. 101 del 2018 si riducono gli alibi di chi non vuole far partire le grandi opere infrastrutturali. Un'altra cosa che chiediamo è di dare continuità agli sconti fiscali per chi investe nel piano impresa 4.0. Il terzo punto è una riforma complessiva dell'aiuto fiscale alle famiglie con figli. Avete voluto un Ministero della famiglia, ma fino ad oggi lo abbiamo visto e sentito poco sul tema delle sue deleghe, se non per annunci sterilmente ideologici. Prevediamo quindi di allargare le tutele a favore dei lavoratori autonomi e degli incapienti IRPEF di inserire un assegno universale di 240 euro mensili per figlio a carico da erogare alle famiglie il cui coniuge con reddito più elevato non superi la soglia dei 100.000 euro annui. quarto ed ultimo punto chiediamo non solo continuità, ma maggiore impegno nello strumento attivo posto a contrasto della povertà: il reddito di inclusione (REI), perché riconosciamo a questo strumento una vera capacità di inclusione attiva e di maggiore incremento verso la partecipazione al mercato del lavoro. Infine, ribadisco il buonsenso delle nostre proposte non aggiuntive, ma sostitutive che - lo ricordo - provano a disegnare un percorso virtuoso di ripresa economica che il nostro Paese per nessun motivo deve smettere di seguire.

la difficoltà di poter comprendere una revisione dell'attuale modello di difesa, che si limita a ridurre le spese militari militari semplicemente con dei tagli in qualche modo immotivati. Altro è un diverso modello di difesa, altro è immaginare dove si può andare a risparmiare, altro è usare la difesa come un bancomat, immaginando che sia una spesa inutile quella di assicurare la sicurezza del nostro Stato e della nostra Nazione, immaginando che si possa azzerare la necessaria previsione a lungo termine che le spese militari prefigurano e rendono necessarie. Per questo motivo voteremo a favore dell'emendamento

di aggiornamento, a riconoscere - attraverso una apposita modifica dell'articolo 119 - il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità

presentazione del provvedimento di iniziativa popolare sull'insularità, ma ritengo che questa iniziativa e questo voto favorevole crei una condizione di giustizia rispetto a quella che è la diseconomia di vivere in un'isola. Chiedo all'Assemblea di leggerlo e interpretarlo;

sul quale la maggioranza di Governo ha votato contro, per cui ciascuno poi si prende le proprie responsabilità.

Signor Presidente, chiaramente il nostro voto è contrario e io approfitto di questi pochi secondi per dare una risposta ad un dubbio

e non riesce a darsi una risposta. C'è la Banca d'Italia, la Banca centrale europea, la Corte dei conti e tanti altri burocrati, investitori e perfino il ministro Savona che ci dice, per tranquillizzarci, se i mercati dovessero continuare ad agitarsi, comunque la manovra potrebbe cambiare. Caro ministro Di Maio, certo, se continua a frequentare ancora il ministro Toninelli, difficilmente riuscirà a darsi una risposta. Questa è una manovra senza obiettivi, confusa, contraddittoria, senza una visione di insieme. È una manovra ricca di egoismo che scarica tutte le responsabilità, tutte le responsabilità sulle future generazioni. Un peso importante. È una manovra che si indebita e con l'indebitamento cosa riesce a fare? Nessun

ma sono luoghi dove si deve incrociare la domanda con l'offerta di lavoro, quindi non è sufficiente il miliardo che voi assegnate ai centri per l'impiego. Quelle risorse serviranno sicuramente per efficientare un sistema che non ma la produzione del lavoro spetta alle imprese. Compito del Governo è facilitare le attività delle imprese e non intralciarle. Avete approvato un decreto-legge chiamato dignità e adesso annunciate la riforma del diritto del lavoro per generare ulteriore confusione e incertezza. Presidente Bagnai,

Sono convinto. Probabilmente voterò a favore, e le spiego perché. Se il Governo sfora il *deficit* con tutte le argomentazioni che lei ha addotto in questa sede,

se lo può fare il Governo, lo può anche il sindaco, che è l'interfaccia dei bisogni primari dei cittadini. Se permettete questo anche ai sindaci, vi assicuro che - in dissenso dal Gruppo del Partito Democratico

che sia garantita la continuità aziendale delle imprese balneari che sono minacciate dalla direttiva Bolkestein. Lo stesso Bolkenstein ha detto che non

del Governo questa necessità ci sembra il minimo. Pertanto, sollecito chi è favorevole a garantire la continuità delle imprese balneari minacciate dalla Bolkenstein a votare a favore dell'emendamento 5.29.

qui sono Maria Teresa, Maria, Luca, Francesco, Giorgio e tanti altri cittadini e cittadine di Roma, in particolare di Villa Spada, Fidene, Colle Salario e Nuovo Salario. costretti a sentire una puzza pazzesca, insopportabile, proveniente dal TMB Salario, impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti. L'impianto è diventato dannoso per le persone in quattro ambiti: ambiente, economia, salute e sociale. Sono quattro ambiti per cui dobbiamo trovare altrettante soluzioni. I TMB erano nati tecnologicamente per ridurre l'inquinamento, perché trattano perché trattano a freddo rifiuti indifferenziati, e per supportare il ciclo virtuoso di riciclo. Ma nell'impianto del Salario ogni giorno vengono portati rifiuti aggiuntivi rispetto a quelli previsti, appoggiati in attesa di essere trasferiti altrove. Quindi, il danno per l'ambiente è che il TMB è stato trasformato in una discarica. La puzza, che è solo il sintomo di questo disequilibrio ambientale, mette a repentaglio la salute fisica e mentale dei cittadini e delle cittadine e la loro socialità. Ero in piazza sabato 6 ottobre accanto alle cittadine e cittadini che manifestavano.

È un danno economico perché in quella realtà le case perdono valore per le famiglie che le hanno acquistate con tanto sacrificio. Il Comune che cosa fa?

parte in causa. La cosa più drammatica è che si fa un monitoraggio non sulle cause della puzza, ma soltanto su quali siano le fonti di calore. Presidente, l'odore è il senso più antico dell'umanità, serve a salvaguardare la vita. Quando un cibo è maleodorante non lo mangiamo; l'odore ci avverte di un incendio. L'odore non ha colore politico. È necessario quindi fare subito un'unità di crisi tra AMA, Regione e Comune e chiudere il TMB Salario, perché le soluzioni per i rifiuti a Roma esistono.

in Sardegna, si stanno ripetendo a livello di uno ogni due o tre anni, talvolta anche un anno dopo l'altro, per cui la parola eccezionale, in questo frangente, non credo sia quella più appropriata. Ringrazio tutti i componenti della Protezione civile, gli assistenti e i volontari che hanno lavorato indefessamente per tutta la notte per ripristinare le condizioni di normalità, cosa che ancora non si è raggiunta nella nostra città. Sono stati provocati danni non indifferenti a tutto il sistema viario e non solo. Si consideri che la raffineria Saras è stata per un certo periodo

i manufatti e le civili abitazioni. Insomma, ogni due o tre anni si ripete la stessa situazione.

Allagamenti diffusi hanno isolato diversi paesi e i Vigili del fuoco hanno dovuto evacuare una sessantina di persone. La viabilità è stata gravemente compromessa. È notizia di pochi minuti fa che una donna dispersa è stata ritrovata morta. Esprimo dunque il mio cordoglio a tutta la famiglia di Tamara, mamma di tre figlie e a tutta la cittadinanza di Assemini. Un ponte è crollato, isolando la strada statale 195, che collega Cagliari a Capoterra. Qualche chilometro prima, un tratto di strada ha ceduto, provocando una voragine, inondata dall'acqua. Altre strade sono state chiuse e così scuole e uffici. Si tratta di zone della Sardegna già duramente colpite dall'alluvione di diversi anni fa. Nel 2008 le vittime furono quattro. Come parlamentare sarda, ma anche a nome di tutti i senatori e deputati, ringrazio tutti i soccorritori e i cittadini volontari che si sono immediatamente attivati; esprimo tutta la mia solidarietà e il cordoglio e auspico che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministro Toninelli mettano in campo tutte le iniziative utili per dare conforto e sostegno alle popolazioni colpite.

famiglie evacuate e ingentissimi danni ai privati e alle attività produttive. Voglio ringraziare, associandomi a quanti l'hanno già fatto, tutta la struttura, gli uomini dello Stato, della Regione e del Comune che sono sul campo, insieme ai volontari, per prestare i primi soccorsi. Questo non è certo il tempo delle polemiche: è il tempo della solidarietà e della vicinanza, ma non è francamente accettabile che si parli di eventi tragici quando sulla strada statale 195 esistono progetti da trent'anni che l'ANAS non porta a compimento. Non è più accettabile che la viabilità rurale, provinciale e quella statale siano in condizioni di abbandono pietoso. da oggi, da qui, parta un'attività intensa, e non solo del Governo e del Ministero, per una ricognizione dello stato di conservazione di queste infrastrutture e per un piano di interventi straordinario, che potrebbe dare risposte anche in termini occupazionali oltre che di sicurezza e di tutela della vita umana.

ai familiari dell'ennesima vittima di situazioni che ormai si ripetono sistematicamente in Sardegna e si portano via delle vite umane. Oggi è mancata una madre di famiglia; c'è ancora

si impiegano due ore e dieci minuti. Purtroppo abbiamo situazioni analoghe, che sono ancora così da cinque anni, da quanto ci fu l'alluvione del 2013. Se non si interviene, vi sono località turistiche che risentono di gravissimi danni, come Cala Gonone, con il famoso ponte di Oloè, di cui tanto si discute, che da cinque anni è bloccato; c'è un ponte sulla Olbia-Tempio

Grazie, Presidente. E proprio qui in Senato, in questo Palazzo di straordinaria bellezza, è stata esposta una sua opera, un olio su tela del 2003, «Il nero e l'azzurro», e mi piace immaginare che questo sia stato d'auspicio e un messaggio per tutti noi parlamentari: vivere la politica, come il maestro ha raffigurato il Mediterraneo, senza angusti confini e orizzonti. Guccione - come ha ricordato l'onorevole Sgarbi in questi giorni - è stato uno dei massimi artisti di livello internazionale per la capacità che ha avuto nelle sue opere di rendere eccezionale l'immagine del Mediterraneo. Dotato di un talento limpidissimo, ha collaborato in giovane età con Renato Guttuso, diventando un punto di riferimento per la sua terra e creando il «Gruppo di Scicli», dov'è nato e dove ha radunato numerosi pittori di cifra realista.

Con il maestro Guccione scompare una delle più alte ed eminenti testimonianze del genio pittorico italiano, che ha onorato non solo la Sicilia, ma il nostro Paese tutto per oltre mezzo secolo. Concludo con una riflessione. Nonostante questo artista abbia vissuto l'intera parabola della vita in una zona depressa, ha saputo trasferirci un messaggio importante. La bellezza esiste dovunque, ma bisogna saperla cogliere e lui, con la sua arte, ha permesso a tutti noi che è possibile scoprirlo in qualsiasi realtà. Grazie, Presidente. Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea su un violento e inaccettabile episodio accaduto il 5 ottobre scorso nei pressi del centro di accoglienza per richiedenti asilo, il CARA di Borgo Mezzanone nel foggiano, dove un controllo stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intense sono le operazioni di contrasto al caporalato in Capitanata, ancor più dopo i tragici incidenti stradali che - come ricorderete - nell'agosto scorso hanno portato alla morte di 16 lavoratori immigrati che viaggiavano su furgoni fatiscenti sulle strade del foggiano.

Da diversi mesi si è intensificato l'impegno nell'attuazione del piano di contrasto al caporalato, viste le condizioni inumane cui sono sottoposti questi lavoratori sia nel lavoro nei campi - tante ore di lavoro a bassa paga - sia nel trasporto in campagna con mezzi sgangherati, sia negli alloggi di fortuna. Nel contempo, è stata avviata una proficua azione di prevenzione e repressione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che ha visto assicurati alla giustizia diversi caporali, alcuni dei quali richiedenti asilo come le loro vittime. È probabile che questi ultimi interventi abbiano acuito l'ira di quegli immigrati che non intendono rispettare le leggi del nostro Stato.

è seguito un inseguimento, anche a piedi, terminato nei pressi del CARA dove il pericoloso automobilista ha tentato di rifugiarsi. Tale CARA è un centro di accoglienza foggiano, è cresciuto a dismisura, diventando una vera e propria zona franca in cui le Forze dell'ordine entrano a proprio rischio e pericolo. Piena solidarietà agli agenti. È doveroso puntualizzare che situazioni simili si sono già verificate e, quindi, ancor più meritorio è l'impegno degli agenti che rischiano la vita con dignità, grande spirito di sacrificio e senso del dovere.

travolse, causando centinaia di evacuati e danni rilevanti. La fragile Italia, per lungo, lunghissimo tempo, è stata trascurata e devastata. Molti fenomeni naturali, seppur pericolosi, per negligenza si trasformano in catastrofi, con vittime e danni enormi. Passando a questi giorni, ricordiamo Stefania Signore con i due figli che, giovedì scorso, in Calabria, è stata travolta e uccisa dalla furia dell'acqua e dell'incuria dell'uomo. Ci addolorano anche le dieci vittime del Raganello. È cronaca di ieri, poi, il nubifragio in Sardegna, già ricordato da altri colleghi. Nubifragi, supercelle e bombe d'acqua sono sempre più estremi e frequenti a causa anche dei cambiamenti climatici. Pertanto, dobbiamo contrastarli globalmente e proteggerci localmente. Non è più tollerabile convivere con rischi naturali da indifesi, a maggior ragione visto che i fenomeni naturali tendono a ripetersi negli stessi luoghi, con le stesse modalità. È giunta l'ora di prevenire tragedie annunciate. Prevenzione deve essere la parola d'ordine anche in quest'Assemblea. Occorre eliminare le cause del rischio idrogeologico e manutenere il territorio. Ogni euro speso sarà un investimento a grande moltiplicatore.

personale, perché quest'oggi in Aula il collega Faraone ha scelto di riferire a suo capriccio le mie parole in Commissione di ieri per poterle ridicolizzare. Ma cosa è accaduto veramente? Lui ebbe a dire - e questo, sì, è successo veramente - che per il reddito di cittadinanza sia stata sacrificata la spesa per la salute degli italiani. A questo ho replicato, e non ad altro, come vorrebbe far passare. Quindi, se la ride e se la canta, ma non ridono gli italiani. Leggo testualmente: «del periodo 2007-2015 la spesa alimentare è diminuita in media del 12,2

non solo meno carne, ma anche meno pesce, frutta e verdura. Così «aumentano i rischi per la salute degli italiani». Non sono parole mie: ne hanno dato notizia ripetutamente gli organi di stampa riportando statistiche ufficiali. E questo gli ho confutato. Innanzitutto, il reddito di cittadinanza non ha sottratto risorse alla spesa sanitaria, che anzi è aumentata nel DEF, ma poi è vero il contrario: insieme alla dignità, il reddito di cittadinanza riporta alle imprese una sospirata ripresa dei consumi interni e alle famiglie italiane restituisce accesso ai farmaci e a una alimentazione più adeguata. Capisco che sia infastidito se le famiglie operaie e i disoccupati vedono restituito, per iniziativa del Movimento, ciò che il PD ha tolto loro di bocca, facendo pagare ai più poveri la crisi e non alle banche. E mi importa anche poco se cerca di burlarsi di me; o se ama storpiare - come è avvenuto - i nomi di Ministri e Sottosegretari. Io non storpierò il suo, ma sulla povertà in quest'Aula non si dovrebbe scherzare.